Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad esprimerci sulla conversione in legge di un decreto-legge che ben prima di essere messo all'ordine del giorno dell'Assemblea ha sollevato un gran polverone nel dibattito pubblico italiano. Infatti le polemiche non sono mancate, e come è giusto che sia per un consesso che rappresenta la volontà popolare, non mancano neanche oggi. Ci sono però alcune cose che mancano, palesemente, e delle quali non sentiamo assolutamente la nostalgia: mancano i risparmiatori disperati, mancano le famiglie straziate dalla consapevolezza di aver perduto tutto ciò che hanno faticosamente accumulato nell'arco della loro vita lavorativa. Ci avete detto che dobbiamo vergognarci perché il Governo populista approva esattamente ciò che era già stato approvato in passato. Cari colleghi, la differenza è sostanziale: oggi non abbiamo una banca con colore politico né una banca in cui si intrecciano legami di parentela familiare tra Ministri del Governo in carica e amministratori presenti o passati della stessa. *(Applausi quando si parla di banche, si ha sempre l'impressione che qualcosa di poco chiaro stia accadendo perché in passato abbiamo vissuto momenti nei quali non si capiva dove finisse la realtà e dove iniziasse la commedia nella vita pubblica italiana. Fortunatamente, ci siamo lasciati alle spalle quei momenti di cui c'è da andare poco orgogliosi. Le tappe fondamentali della vicenda Carige le conosciamo tutti: molti avevano capito da tempo che la situazione era irrisolvibile, altri lo hanno capito a novembre quando l'istituto non è riuscito a vendere sul mercato un *bond* subordinato e per questo si è reso necessario l'intervento del sistema bancario con 320 milioni versati in Carige dallo schema volontario del Fondo interbancario. Le tappe, ripeto, le conosciamo tutti, così come sappiamo che i capisaldi del decreto-legge - cioè la garanzia, l'intervento dello Stato e la condivisione degli oneri sono le azioni immediate più efficaci che il sistema di norme europee nel quale siamo inseriti ci consente di attuare velocemente, allontanando lo spettro del *bail in* che tanto male ha fatto ai nostri risparmiatori. E proprio la rapidità con la quale il Governo è intervenuto, emanando il decreto-legge a stretto giro dopo il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato dalla Banca centrale europea, ed in sostanziale continuità con esso, ha permesso la tutela sia del risparmio che dei posti di lavoro degli impiegati di Carige, che ammontano a ben 4.200 unità. Il nostro sistema bancario va tutelato, su questo siamo tutti d'accordo, e va sostenuto perché senza un sistema bancario nazionale forte, radicato sul territorio e capace di fornire sostegno all'attività di imprese e famiglie, rischiamo di perdere uno

non fosse intervenuto avremmo perso quel legame fecondo che esiste tra Carige ed il territorio della Liguria. Un legame sul quale la fiducia dei nuclei produttivi liguri deve tornare a costruire benessere e produttività, e per farlo c'è bisogno di un ritorno della banca ad uno stato di salute sufficiente da meritare quella fiducia senza la quale è impossibile la ripartenza. Certamente, Presidente, il decreto-legge è soltanto uno strumento e abbiamo visto quanto sia stato usato male in passato, per tutelare i banchieri anziché i risparmiatori. ha raggiunto un tasso di sofferenza tale da indurre le istituzioni a intervenire, qualcuno ne è colpevole e deve pagare un conto salato: ne va della nostra stessa funzione di rappresentanza della volontà popolare. come sia possibile che ancora una volta una gestione spericolata e avventata delle risorse di una banca, l'utilizzo di prestiti su cui è calata l'ombra del sistema clientelare e un'opera costante di investimenti in settori spesso sbagliati abbiano potuto perpetuarsi per anni, nonostante esistano precise realtà deputate alla vigilanza bancaria. Dobbiamo, ancora una volta, chiedere conto del perché non è stato possibile evitare l'ennesimo tracollo di una banca strategica per l'economia locale e nazionale.

degli italiani deve pagare due volte. Da ligure e rappresentante dei cittadini liguri, saluto questo provvedimento con soddisfazione e torno a casa a testa alta perché i cittadini sanno bene che, nonostante ciò che dicono le opposizioni, noi siamo molto diversi da quanti e M5S).* Del resto basta chiedere alle associazioni dei risparmiatori truffati da Banca Etruria e dalle banche venete, per i cui risarcimenti in manovra di bilancio sono stati stanziati 1,3 milioni di euro, se avrebbero preferito nei loro casi avere a che fare con la celerità e la serietà di questo Governo oppure no. La risposta è stata già data alle urne dello scorso anno. *(Applausi

da cittadina ligure vivo con particolare coinvolgimento il caso di Banca Carige e se intervengo in questa sede, per parlare del decreto-legge del nostro Esecutivo, che stiamo convertendo in legge, è perché sono convinta che ciò che stiamo facendo come Governo sia la cosa migliore da fare, prima di tutto per i cittadini, liguri e di tutta Italia. Il provvedimento è un intervento a sostegno di una banca totalmente diverso da quelli del Governo che ci ha preceduto, perché è tempestivo e non c'è alcun regalo ai banchieri: il capitale versato dallo Stato, in garanzia delle emissioni obbligazionarie dell'istituto, dovrà essere restituito. Inoltre, per tutta la durata dell'intervento statale, la banca non potrà distribuire dividendi. Siamo dunque, ancora una volta, ad intervenire con urgenza sulla crisi di una banca.

Il nostro Governo, nella manovra, ha messo un miliardo e mezzo di euro per aiutare gli azionisti truffati dalle banche. Cifra, mi piace far notare, 15 volte superiore all'elemosina di 100 milioni che era stata prevista dal Governo Gentiloni Oggi, ancora una volta, ci troviamo a riparare i danni che voi avete fatto chiudendo gli occhi di fronte a una gestione vergognosa delle banche, della vigilanza e delle crisi in generale. C'è un'altra novità rispetto al passato, che mi rende orgogliosa della legge di cui stiamo discutendo oggi. Grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle, a firma Currò, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetterà al Parlamento una relazione ogni quattro mesi per rendere pubblici i debitori di un certo peso della banca ligure e per far capire tempestivamente quali e quanti crediti dell'istituto rischiano di andare in sofferenza. Ricordo la mia reazione quando ho letto i nomi di chi, avendo ricevuto prestiti facili senza restituirli o facendolo solo in parte, con la complicità dei dirigenti, ha affossato la banca. Rimasi indignata e, dopo aver letto quei nomi, la reazione dell'opinione pubblica è stata la stessa. Nomi noti a noi liguri e non solo, perché non si tratta di gente comune, ma delle *élite* della cosiddetta imprenditoria, della politica e della società, in Regione e non solo. Finalmente questi nomi non sono coperti dalla politica, queste persone non sono protette da un Governo compiacente. Come abbiamo già fatto e come continueremo a fare grazie a questo emendamento, scoperchieremo i legami tra le banche e la politica; legami che, anche nel recente passato, hanno funestato la gestione di Carige. Sapete perché questo mi fa indignare? Perché se da questa parte abbiamo i soliti noti, dall'altra parte ci sono milioni di persone comuni in Italia che non hanno né "santi in paradiso", né amici negli istituti bancari, ai quali non viene prestato nemmeno un euro dalle banche, sia che si tratti di fare impresa, sia che si tratti di necessità del momento. I costi della crisi sono stati riversati dalle banche sui loro clienti e si sono tradotti in prestiti più onerosi e restrizioni del credito. La nostra economia era fondata proprio sul credito bancario e questo scenario è una delle principali cause della più grande crisi del dopoguerra, quella del decennio 2007-2017,

Oggi in Italia stiamo cercando di risolvere, dunque, vecchi problemi, ma cerchiamo di farlo con soluzioni nuove, visto il fallimento di chi ci ha preceduti e che oggi vorrebbe darci lezioni. Il decreto-legge approvato nel Consiglio dei ministri del 7 gennaio scorso che oggi esaminiamo ha lo scopo di proteggere in via precauzionale i risparmiatori. Offriamo una garanzia fino ad un massimo di 300 milioni sui prestiti ottenuti da Banca Carige, che siano raccolti sul mercato o da Banca d'Italia. Come accennato, nel caso in cui la banca non dovesse riuscire a restituirli, interverrà lo Stato; in questo modo per Carige sarà più facile raccogliere liquidità e garantire l'operatività della banca. Solo nell'ipotesi in cui Banca Carige non riuscisse ad adeguare i suoi requisiti patrimoniali, anche attraverso un accorpamento, lo Stato interverrà direttamente ricapitalizzando e garantendo correntisti e risparmiatori. In questo caso però, sia ben chiaro, la banca diventerebbe di proprietà pubblica, cioè dei cittadini stessi, e non regaleremo questa banca, come è stato fatto in passato, ad un'altra banca privata per la cifra simbolica di un euro facendo pagare il conto ai risparmiatori. Il messaggio deve essere chiaro per tutti: con noi è finita l'era dei profitti privati fatti coi soldi pubblici. Gli italiani, esattamente un anno fa, ci hanno chiesto di cambiare il modo di fare politica; ci hanno chiesto di farlo concretamente, non solo a parole, e il provvedimento in discussione è la prova provata che manteniamo la parola data, perché se è vero che abbiamo ereditato un sistema Paese in macerie, è altrettanto vero che non ci stancheremo mai di rimediare ai danni fatti, di ricostruire un Paese sulle fondamenta solide dell'etica e della dignità

ritengo sia certamente condivisibile, ragionevole e opportuno per le misure di tutela che propone agli amministratori straordinari di Banca Carige e per metterli in grado di operare al meglio al fine di riuscire a risollevare le sorti dell'Istituto dopo il destino

le responsabilità che nel corso degli anni si sono accavallate; la magistratura sta procedendo penalmente nei confronti degli ex vertici di Banca Carige per i reati noti e vedremo se l'accertamento della responsabilità penale contribuirà a far luce su quelle che già oggi, prima ancora di alcune sentenze, appaiono come le solite musiche italiane di vicinanze del potere economico, finanziario, bancario a gruppi di potere e troppo spesso al potere politico. A parte questo,

operazioni di verifica, questi *stress test* che, come sappiamo, sono dei procedimenti mediante i quali le banche sono sottoposte a simulazioni rispetto a cosiddetti scenari avversi per verificarne la solidità,

è una società di investimenti che svolge consulenza anche alle banche private, oltre che ai Governi e agli Stati, che devono rispettare i requisiti imposti dagli stessi *stress test*. Sto evidentemente facendo riferimento a una situazione di conflitto di interessi che a me pare grande quanto una cattedrale. *(Applausi che svolge legittimamente il suo ruolo fra i principali *player* mondiali del mercato finanziario, della gestione dei crediti deteriorati, delle partecipazioni azionarie, della partecipazione nei consigli di amministrazioni di società di mezzo mondo? Faccio presente che BlackRock, una società americana, naturalmente, con sede a New York, gestisce direttamente un patrimonio di 6.300 miliardi di dollari. Cifra che qualcuno si è divertito a paragonare al PIL di intere Nazioni come Francia e Spagna, nel suo insieme. Gestisce, indirettamente, mediante partecipazioni azionarie in società che sono dappertutto, il settore finanziario, dei trasporti, dell'energia.

circa 20.000 miliardi di dollari. Ripeto: 20.000 miliardi di dollari. Quindi, è un colosso. Probabilmente, è uno dei padroni del mondo. dei *player* che, in campo globale, agisce, verosimilmente, determinando le sorti, non solo di banche piccole o grandi, ma di intere Nazioni. E io di questo non ne faccio una colpa. Non sto additando BlackRock come fosse il diavolo, perché nel sistema economico in cui siamo immersi, ultracapitalistico,

le operazioni di *stress test* di un gruppo di banche, tra cui anche Banca Carige, nel 2018 (i cui esiti mi pare siano stati pubblicati alla fine dello scorso anno), io anno), io chiedo a chi ne sa più di me se questo, magari, possa avere influito sulle vicissitudini che hanno interessato Banca Carige proprio nell'ultima parte dell'anno. Sappiamo che l'assemblea straordinaria del 22 dicembre ha visto le dimissioni degli amministratori, con tutto quello che è accaduto nelle settimane successive, e l'intervento tempestivo e provvidenziale, secondo me, del Governo, che ha proposto il decreto-legge in esame. BlackRock non si limita a fare consulenza

agisce anche nel mercato degli NPL, dei *non performing loan*, dei crediti deteriorati. Sappiamo che nel piano di ristrutturazione proposto dagli

non esigibili o di difficile esigibilità. È il caso di considerare che BlackRock, sebbene non sia certamente l'unica, è una delle più grandi società che in ambito planetario si muovono anche nella gestione di questo tipo di crediti deteriorati. tratta di circostanze certamente già note agli operatori del settore; non dico nulla di nuovo: la stampa specializzata italiana nel mese di dicembre - «Il Sole 24 Ore», ad esempio - ha rilevato questa situazione. Ho visto che altri colleghi,

ha interloquito con l'autorità bancaria europea per chiedere lumi e spiegazioni su questa circostanza invero astrusa, che fa trasparire un conflitto di interessi francamente, anche un bambino di sei anni potrebbe riscontrare. Abbiamo quindi avuto le risposte da parte del Presidente della Banca centrale europea, che si occupa di verificare gli scenari bancari e

l'esame dei bilanci delle banche al fine di trarne vantaggio. Ebbene, credo che bisogna essere forse un po' ingenui, o troppo buoni, se ci si aspetta che società, che fanno legittimamente del profitto sui mercati finanziari,

in Italia, Paese che forse più di altri sta soffrendo le politiche monetarie e finanziarie da parte della BCE, dobbiamo stare zitti? Non è forse questa una grande occasione

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame comporta misure urgenti a sostegno di Carige, la Cassa di risparmio di Genova e Imperia, conseguenti alla bocciatura dello stato patrimoniale, derivata derivata dall'azione del Meccanismo di vigilanza unico europeo e dalla decisione degli azionisti di non procedere, nell'assemblea di dicembre, all'aumento di capitale. Un provvedimento con il quale

Si tratta di un intervento inevitabile, inevitabile, esattamente come inevitabili furono gli interventi a sostegno delle Banche venete e di Monte dei Paschi di Siena. I focolai di crisi vanno spenti prima che si determinino squilibri finanziari del sistema bancario. Carige è una banca solvibile, come è stato detto prima, con oltre 500 sportelli bancari, 4.200 dipendenti, un milione di clienti. Va quindi ristabilito un clima di fiducia. Infatti, solo così potrà essere preservata l'erogazione del credito all'economia reale e, quindi, mantenere l'occupazione ed evitare l'appesantimento del nostro debito pubblico. Sicuramente, come abbiamo

a quello che venne approvato nel 2016 dal Governo di centrosinistra. Non è un fattore di poco conto, perché intorno a quel provvedimento venne costruita una demagogica campagna di attacco al Governo di centrosinistra.

dei loro atteggiamenti istituzionali di allora. Non esiste una contrapposizione politica su questi temi. Le banche sistemiche vanno salvate per evitare che l'economia crolli e salvare gli aspetti che caratterizzano l'economia reale, soprattutto i posti di lavoro. Si tratta di un concetto che dovrebbe valere sempre e non diventare mai materia di contesa elettorale. Sarebbe utile capire ora quale deve essere il futuro di Carige. Il Ministro, nell'audizione presso le Commissioni congiunte di Camera e Senato, ha auspicato una soluzione di mercato. Il vice *premier* Di Maio ha invece più volte elogiato i vantaggi di una banca di Stato. Credo che, alla luce Paese, le banche commerciali di Stato non hanno certo brillato per efficienza o etica. La nazionalizzazione deve essere l'ultima istanza e, comunque, temporanea. Ritengo che per dare un futuro a Carige bisogna fare un'analisi chiara della situazione italiana. Molti istituti si stanno sottraendo e appaiono sempre meno interessati ad acquistare Carige. Soprattutto, per incentivare l'aggregazione, che può essere una via di uscita, bisogna isolare la mole di crediti deteriorati, che è ancora un problema rilevante. In questo senso, come previsto nelle proposte migliorative che

sostenere la Società per la gestione di attività - la SGA - che è l'intermediario finanziario che si occupa del recupero dei crediti deteriorati. La stabilità finanziaria è una condizione necessaria per la tutela del risparmio.

la certezza di essere rimborsati per coloro che sottoscrivono obbligazioni o azioni senza una piena comprensione dei rischi. Inoltre, c'è un aspetto non secondario e molto rilevante, che è il completamento dell'unione bancaria. A mio avviso, c'è una contraddizione forte tra la supervisione e le decisioni sulla gestione delle crisi, che ha una connotazione europea,

L'obiettivo deve essere costruire un sistema che garantisca la stessa tutela ai risparmiatori di tutta Europa. Solo così potrà essere reciso il circolo vizioso tra crisi bancarie e crisi del debito sovrano. Solo così potremo affrontare le crisi giocando d'anticipo. Per questo credo sia stato sbagliato l'atteggiamento di attacco a Bankitalia e alla Consob che avete promosso negli ultimi mesi, soprattutto in un periodo di grande volatilità finanziaria dei mercati. Io credo che il miglior obiettivo che ci dobbiamo dare sia garantire a questo Paese un percorso di crescita. È fondamentale che, parallelamente all'attenzione ai problemi finanziari e alla cura della stabilità finanziaria, ci sia una strategia di crescita importante. Noi ci troveremo nei prossimi mesi di fronte a un cambiamento di scenario. un aspetto fondamentale, che è la conclusione del sostegno della Banca centrale europea al nostro sistema bancario bancario (con il *quantitative easing* che termina). A giugno le nostre banche dovranno ricominciare a ripagare gli strumenti di liquidità offerti dalla Banca centrale. Lo *spread* è costantemente più alto della media europea. Credo che con la recessione, con i dati che abbiamo e che caratterizzeranno il 2019, si correrà il rischio di aumento delle sofferenze. Secondo me dobbiamo allora impegnarci - e lo dovete fare soprattutto voi che siete al Governo - verso una strategia di crescita, abbandonare la politica di decrescita ostile agli investimenti e dovete impegnarvi a rilanciare le infrastrutture e una politica per l'attuazione dell'unione bancaria. Abbiamo bisogno di scelte e non di recriminazioni. Abbiamo bisogno di guardare al futuro e non di cercare i capri espiatori. C'è bisogno di un periodo in cui tornino a primeggiare l'etica della responsabilità e soprattutto la centralità della responsabilità della decisione. Non è più possibile continuare sulla ricerca dei capri espiatori: è sempre colpa di qualcun altro, una volta dell'Europa, una volta di quelli che c'erano prima. È una strada sbagliata. Noi voteremo il provvedimento in esame con convinzione a patto che il tema in questione non diventi più un elemento demagogico di contesa elettorale.

Italia. Siamo d'accordo rispetto al decreto-legge, perché lo siamo sempre stati: siamo sempre stati favorevoli a risolvere e a stabilizzare le crisi del sistema bancario, perché esso è interdipendente. Senza un sistema bancario solido, non ci sono famiglie, non ci sono cittadini, non ci sono imprese, non c'è crescita economica e sociale nel Paese. Pertanto, le sciocchezze che sono state dette rispetto a questo decreto-legge,

e solo se - il sistema bancario è solido. Questo va detto perché è un principio fondamentale. Non ammettiamo più di sentire sciocchezze che mettono in discussione i pilastri fondamentali della nostra Costituzione.

instabilità. Abbiamo sentito parole molto costruttive - anche ieri dalla commissaria Vestager - in quest'Aula. Abbiamo sentito che si può e si vuole modificare il *bail in*; che si può diluire la normativa sugli NPL; che si vuole andare verso la costruzione di un sistema bancario unitario, che guardi non solo alla vigilanza europea, ma anche a una stabilizzazione unitaria europea. Ma come si può costruire tutto questo continuando a fare polemica con tutti in Europa, con tutti gli Stati? È un atteggiamento insopportabile, a parte il fatto che va davvero nella direzione opposta rispetto a quella unica utile all'Italia. politica, abbiamo sentito delle *boutade* assurde, che hanno fatto schizzare lo *spread* e hanno fatto perdere 300 miliardi al sistema Italia. La capitalizzazione delle banche è calata drasticamente,

giusto per dare l'idea dell'immensità di tali sciocchezze: è stato detto che si potevano non restituire 250 miliardi di prestiti alla BCE, oppure che c'era un piano B per uscire dall'euro. Sono affermazioni dannosissime. forte. Se tutto questo fa male alle banche *in bonis*, fa ancora peggio alle banche che, come Banca Carige, da anni soffrivano ed erano in difficoltà.

un proseguimento dei *talk show* o un luogo dove fare inquisizione sulle responsabilità del passato. Non spetta alla politica fare inquisizione, ma spetta alla magistratura appurare le responsabilità.

e imporre nomine discutibili in termini di indipendenza rispetto alla Consob. Banca d'Italia e Consob sono agenzie indipendenti, a garanzia del sistema, a garanzia degli investitori, a garanzia dei risparmiatori, e quindi non è tollerabile, in base alla Costituzione e per l'Italia che noi conosciamo, questo tipo di ingerenze della politica. Questo non è costruttivo: è un atteggiamento che ha messo fortemente in discussione un sistema bancario che andava ripensato con grande lungimiranza.

alle regole che tutti conosciamo e che il Governo conosce sugli aiuti di Stato, perché crea un'ingiustificata concorrenza tra banche, com'è naturale. Perché, allora, non si sono volute adottare soluzioni molto più ragionevoli, come avere dei lodi certi dell'arbitrato Consob? Volevate

quello per un'Italia che deve essere vista come un sistema unitario e interdipendente. Non esiste dicotomia tra lavoratori e imprese; non esiste dicotomia tra risparmiatori e banche e non esiste un Governo che possa stare in maggioranza e possa dirigere il Paese che non abbia chiaro che lavorare per i cittadini è lavorare a favore di un sistema interdipendente. Quello che abbiamo sentito fino ad oggi, un costante essere contro, è il ruolo di una forza di opposizione. Se non siete in grado di governare il Paese, fate quello che siete capaci di fare: tornate all'opposizione. Noi votiamo Carige.

La causa è da attribuire *in primis* alla crisi economica. A fronte delle difficoltà delle famiglie e delle imprese a far fronte ai debiti contratti con le banche, le stesse hanno prodotto crediti deteriorati, deteriorati, che, tra il 2013 e il 2015, sono cresciuti in maniera esponenziale nel bilancio delle banche, fino a diventare esplosivi. Le perdite accumulate di anno in anno hanno finito per portare il patrimonio di alcune banche a livelli tali da non garantire più la loro solidità. È quello che è successo alle banche venete, a MPS, alle barche del Centro Italia, come Banca Etruria, e oggi a Banca Carige. Ma «le banche italiane sono solide», diceva fino a un anno fa l'ex *Premier*, oggi collega, Matteo Renzi. Ma vi è di più. Non possiamo nasconderci che un'altra causa della crisi del sistema creditizio è da attribuire a gravissimi errori gestionali e amministrativi della *governance*; caso anche la politica dei passati Governi non è esente da responsabilità. Difatti, l'intreccio tra politica e banche è noto a tutti: prestiti concessi a grossi imprenditori, amici degli amici, i quali non li hanno restituiti, creando appunto quei crediti deteriorati che poi hanno portato al fallimento di alcuni istituti di credito. Con l'introduzione della direttiva comunitaria n. 59 del 2014, cosiddetta di risoluzione delle crisi bancarie, entrata in vigore nel 2016, si è introdotto un principio secondo cui lo Stato non deve più farsi carico del salvataggio dell'istituto di credito in crisi. Se una banca fallisce, i primi a essere chiamati in causa devono essere gli azionisti, poi gli obbligazionisti e solo alla fine i correntisti con depositi sopra i 100.000 euro, mentre sotto i 100.000 euro sono garantiti da un fondo interbancario. Si chiama salvataggio interno, in inglese *bail in*. C'è una terza via, prevista sempre dalla direttiva europea, per salvare un istituto di credito: la ricapitalizzazione precauzionale ad opera dello Stato; di fatto una nazionalizzazione, che può essere fatta però solo ad alcune condizioni. Ebbene, questa è una delle misure previste dal decreto-legge n. 1 del 2019, recante misure urgenti di sostegno alla Banca Carige e ai suoi risparmiatori, che oggi siamo chiamati a convertire in legge, insieme alla copertura delle emissioni obbligazionarie di Carige: una copertura ammessa dall'ordinamento comunitario.

2019, dopo il cambio di ben quattro amministratori delegati e tre presidenti in soli tre anni; fatto che non ha consentito quelle importanti iniziative di riassetto che sarebbero state necessarie a fronte di circa 3,5 miliardi di crediti deteriorati. Ebbene, con estrema urgenza e necessità il Governo giallo-verde è dovuto intervenire al fine di mettere in sicurezza la banca, ma soprattutto i risparmiatori, con una disciplina che al momento non ha comportato alcun esborso per lo Stato e, quindi, per i cittadini italiani. Si tratta di 1,3 miliardi, stanziati per permettere alla Banca Carige di stare sul mercato e risollevarsi, ma soprattutto per evitare il *bail in*. Sono soldi pubblici che non sono ancora usciti dalle casse dello Stato e che si spera non usciranno mai. Anzi, al momento questa garanzia è risultata onerosa per l'istituto. Il salvataggio interno, cosiddetto *bail in*, sarà dunque l'*extrema ratio* per questo Governo. Si tratta pertanto di un'operazione diversa da quella fatta dal Governo Renzi, che prima ha ratificato il *bail in*, poi lo ha applicato e infine, solo dopo aver visto il grosso danno fatto ai risparmiatori, è intervenuto con un investimento pubblico di ben 20 miliardi

tanto da lasciare in terra tanti risparmiatori, che noi del Governo giallo-verde abbiamo dovuto risarcire con uno stanziamento di un miliardo e mezzo di euro. Dunque, non c'è alcuna contraddizione del MoVimento 5 Stelle quando dice che lo Stato non deve salvare le banche, perché la predisposizione di garanzie pubbliche alla risolvibilità di Carige è stata dettata proprio dalla necessità

a nostro parere - contrasta con la Costituzione e, precisamente, con quanto disposto dall'articolo 47 sulla tutela del risparmio. Quindi, l'intervento preventivo del Governo giallo-verde, nel caso di Carige, per evitare il *bail in* è più che giusto.

è stata contestata quando era il momento di inserirla nell'ordinamento giuridico italiano? Dopo il recepimento, infatti, si è passato il tempo a cercare di non far scattare il *bail in*. Lo stesso governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco invitò l'allora Governo Renzi ad avviare una revisione della direttiva UE, ma niente è cambiato da allora e la legge è rimasta quella. Tante sono le direttive comunitarie che l'Italia non applica, seppure pagando sanzioni che oggi - possiamo dire - ci sarebbero costate molto meno di tutti i miliardi spesi finora per salvare i risparmiatori, con danni invece irreparabili alla fiducia nelle banche da parte dei

a fronte di affermazioni del tipo: «Non accettiamo *Diktat* della Commissione europea», viene seguito esattamente il percorso che la Commissione europea ha imposto E il percorso prevede una serie di passaggi, finiti i quali entra la ricapitalizzazione precauzionale dello Stato, cioè il *burden sharing*, la condivisione dei dei fardelli. Ciò vuol dire che verranno azzerati nell'ordine gli azionisti, gli obbligazionisti *junior* e gli obbligazionisti *senior.* Ci sarà il solito bagno di sangue a cui abbiamo già assistito con Banca Monte dei Paschi di Siena.

fresco per una nuova ricapitalizzazione. Quando l'azionista di riferimento - in questo caso la famiglia Malacalza - dice di non avere più soldi o di non volerne più tirare fuori se non si capisce dove vuole arrivare la banca, è chiaro che a quel punto si deve intervenire. Il momento è quello: non è né prima, né dopo. Non lo sceglie la politica: lo scelgono

il fatto che lo Stato entri nel capitale azionario non vuol dire che la banca viene nazionalizzata. La banca viene nazionalizzata solo nel momento in cui lo Stato fa un'OPA residuale delle azioni che mancano

non rende più nulla da tanti anni. Questa è la vera questione alla quale bisogna puntare: visto che prestare soldi non rende, le banche hanno dovuto trovare altri sistemi per impiegare l'enorme massa di risparmio che la collettività ci ha riversato dentro con strumenti finanziari a più alta resa.

È troppo rapido il modo in cui vengono bruciati i soldi: vuol dire che ci sono strumenti finanziari a leva, derivati di copertura o non di copertura, quotati oppure fuori dai mercati regolamentati, che causano un'erosione del patrimonio colossale.

oltre alla necessaria separazione tra attività di banca tradizionale e attività di banca d'affari, bisogna anche mettere un freno a quello che può fare una banca d'affari. È dal 1997,

l'esplosione del sottostante causa un'esplosione praticamente immediata del derivato. Su questo il Governo sta facendo qualcosa? Nella scorsa legislatura c'erano tanti progetti di quella che allora era l'opposizione per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali e per un certo tipo di regolamentazione. Questo è il pilastro fondamentale sul quale ci si dovrebbe muovere, altrimenti Banca Carige sarà solo una delle tante banche che hanno problemi finanziari. Non faccio nomi, ma chiunque avesse voglia di andare a guardare il conto economico di altre banche vedrebbe che quelle in difficoltà sono abbastanza. Finché sono banche di media dimensione il sistema può tollerarlo, ma fino a che punto si può accettare un'immissione di liquidità nel sistema bancario per tutelarne la stabilità? Ci sono banche più grandi, per le quali gli ultimi aumenti di capitale sono stati superiori ai 10 miliardi di euro, che non possono ragionevolmente sopportare un ulteriore aumento di di capitale in caso di erosione del patrimonio di vigilanza. Tutte queste sono domande alle quali bisogna dare risposta, prima che i mercati diano risposta al posto nostro. Un'ultima considerazione - e concludo - relativamente al *bail in*: la

questo decreto-legge. Fratelli d'Italia non è d'accordo su questa passiva acquiescenza, ma vorrebbe cercare, almeno in alcuni particolari, di portarvi un contributo costruttivo. Mi rivolgo

Sempre nel merito e nella tecnicità di questo mio intervento, che cosa vogliamo dire del fatto che il pubblico andrà a salvare e a beneficiare un'azienda privata, una banca,

i *bonus*, i compensi e gli extra compensi dei *manager*, magari tenendo conto della linea del pubblico impiego, avrebbe allora un senso nel momento in cui si chiede alla mano pubblica di intervenire in questo contesto. Anche qui, amici a cinque stelle, vi sfido sulla coerenza con il vostro passato.

che su questo sistema venga fatta chiarezza, che non vengano utilizzati per politiche di bilancio né svenduti per poi arricchire qualche gruppo finanziario. Soprattutto, sempre a proposito di NPL, proponiamo anche un emendamento nel semplice interesse del debitore onesto perché, se ci sono stati - e sicuramente ci saranno

noi chiediamo allora che per le piccole imprese e per i cittadini sia possibile riacquistarli, con una piccola integrazione, dal cessionario. È un'esigenza di onestà e di chiarezza nei confronti dei nostri piccoli imprenditori e dei nostri cittadini risparmiatori, che vedono invece spesso lucrare alle proprie spalle, per poi ritrovarsi la necessità di pagare interamente quel debito che la banca ha ceduto all'8, al 10, al 12 per cento del suo valore.

aiutandomi con la citazione dell'ultimo sforzo editoriale del ministro Savona, ministro in carica, candidato alla Presidenza della Consob; un candidato discusso, probabilmente non discutibile.

alcune domande: serviva il decreto-legge Carige? In quali termini? Serviva esattamente in questo momento? C'è un'alternativa? Ci sono stati dei precedenti?

soprattutto nell'ultima legislatura, quella prima dell'attuale, per la quale avrei voluto essere presente, perché il poter dire adesso su questo argomento, se avessi potuto contare sull'esperienza da spettatore, sull'incendio della ragione dell'ultima legislatura, sarei stato di sicuro più efficace, più convincente, più capace anche di comunicazione immaginifica. Ora non voglio realizzare l'incendio della ragione. Voglio dire che non c'era altra iniziativa che quella che è stata assunta. È per questo che i Gruppi parlamentari voteranno, per la maggior parte, a favore, totalmente convergenti salvo alcuni distinguo, che però produrranno un voto di responsabilità. Sappiamo infatti che Banca Carige non è esattamente un elemento di abbellimento della città di Genova: Banca Carige è una delle infrastrutture grazie alle quali si dovrà rideterminare la ripresa del volo, del largo della città di Genova, dopo la vicenda del ponte Morandi, che non ha riguardato soltanto un ponte, ma ha rappresentato proprio la caduta di fiducia nel futuro. Banca Carige ha avuto sofferenze e difficoltà. Noi abbiamo sentito tre autorità in Commissione: il ministro Tria, il vice direttore generale Panetta - leggo questa mattina, candidato alla direzione generale - e il vicariato innominabile di Consob.

onerosamente per precauzione, sulla finanza pubblica; ma, per completare il cammino, servirà che il mercato si faccia carico della rigenerazione di questa banca. Si è sbagliato quando si è detto, da parte di figure che hanno un ruolo di Governo in questa maggioranza, che la via d'uscita sarebbe stata la nazionalizzazione. Si parla a caso, se si parla in questi termini. Noi dobbiamo fare in modo che il mercato produca la soluzione, sapendo che la normativa può essere anche di facilitazione - ad esempio - sul piano fiscale, come ci hanno suggerito gli auditi in Commissione: lavorare su una normazione che faciliti, dal punto di vista fiscale, procedimenti di riaggregazione, di ingrandimento e ristrutturazione.

per fare in modo che non ci siano più quelle debolezze pagate e patite in passato. Dobbiamo fare in modo - ad esempio - che coloro i quali hanno patito la sfortuna di una banca che ha conosciuto sfortuna, i risparmiatori, siano risarciti, evitando, però, che la norma sul risarcimento venga saccheggiata dalla politica. Anche questo è stato detto dal ministro Tria in audizione. Il concepito normativo del Governo funzionava; poi il Parlamento l'ha saccheggiato, per ragioni elettorali, e adesso c'è una fase di stanca, c'è la palude, tant'è che anche la commissaria Vestager è venuta a ripeterci che vi sono difficoltà sulla procedura da attivare per quanto riguarda il ristoro dei risparmiatori traditi. Cosa serve allora? Evitiamo di metterci la polemica politica, la lettura ideologica. Evitiamo di incendiare la ragione, quando trattiamo di istituzioni fondamentali per l'economia, per la società e per il futuro. Giorgio Ruffolo diceva che non sempre il denaro depositato è lo sterco del diavolo: quando il denaro depositato è funzionale a progetti di vita, di ambizione delle imprese e del territorio, esso diventa molla, funzione. Sappiamo che è per questa ragione che la Costituzione ha stabilito, all'articolo 47, la tutela del risparmio, la sua custodia rispettosa, la sua protezione e, dall'altra parte, il controllo dell'uso del credito. Su questa base,

È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà. Presidente, colleghi senatori, oggi siamo qui in Aula per votare un provvedimento che mai avremmo

quando si sostituisce alla comprensione. Questo discorso però non ci appassiona più di tanto; non si tratta di puntare il dito contro chi fa queste inversioni e fa retromarcia su tutti gli argomenti; a noi interessa

clausola inserita nella legge di bilancio oggi siete riusciti a bloccare. In due anni si erano raccolti 23 miliardi di euro di risparmio privato. In cinque anni, con quelle che erano le agevolazioni fiscali, si sarebbero raccolti 150 miliardi di euro, che andavano a finanziare l'economia reale del Paese. Siete stati capaci di bloccare anche questi strumenti! Siete capaci, oggi, di combinarne veramente tutte! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Come dicevo, questo provvedimento si limita oggi ad affrontare il caso Carige. Lo avete fatto con il copia-incolla di un decreto, che è quello passato, il tanto criticato decreto Gentiloni Silveri sul Monte dei Paschi di Siena. Non si prevede assolutamente, oggi, quella che è una riforma importante, proprio di sicurezza del settore bancario e di tutela del risparmio degli italiani. italiani. Per andare verso la conclusione del mio intervento, vorrei citare alcuni dati di quello che è oggi il sistema bancario italiano, molto forte, molto importante e molto strutturato del nostro Paese. In Italia noi abbiamo 538 banche attive.

ha perso circa 44.000 posti di lavoro. Gli occupati del sistema bancario sono scesi da 330.000 a 286.000. Nel 2008 anche il numero degli sportelli, che sono importanti sul nostro territorio, al servizio dei cittadini, è diminuito del 20 per cento. L'emorragia - ahimè - dei posti di lavoro continuerà, perché ci sono piani di uscita, soprattutto dei grandi gruppi bancari. Al Nord si è perso un addetto ogni dieci. Al Sud si sono persi due addetti ogni dieci del sistema bancario. È un tributo occupazionale enorme, che dobbiamo cercare di evitare a tutti i costi, perché dentro il mondo bancario ci sono anche famiglie, cittadini, uomini e donne che lavorano per il nostro Paese.

Il nostro sistema bancario ha prodotto circa il 5,7 per cento del PIL nazionale, secondo soltanto al Regno Unito, e primo rispetto a Francia e Germania che hanno prodotto il 4,5 e il 4,1 per cento. Quindi, un sistema bancario solido, un sistema bancario forte, che, come dicevo, non soltanto oggi deve necessariamente tutelare i risparmiatori italiani, ma che genera anche prodotto interno lordo. Quindi, necessariamente dobbiamo guardarlo con fiducia e dobbiamo intervenire con fiducia nel settore. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, ricordando a tutti come Forza Italia

il ruolo delle banche come Banca Carige, che sono un patrimonio assolutamente importante del nostro sistema, un patrimonio fondamentale per il tessuto economico del nostro Paese.

signori rappresentanti del Governo, le garanzie pubbliche per salvare Carige, una strada obbligata dettata dalla necessità politica di scongiurare l'attivazione del *bail in*,

solo dopo che le risorse interne, compresi i conti correnti oltre i 100.000 euro ed i *bond* subordinati, siano state drenate per ripianare parte delle perdite dell'istituto in crisi. Norma che contrasta palesemente con l'articolo 47 della Costituzione. Qualche giorno fa, ad una mia domanda in Commissione finanze del Senato su questa direttiva, che è stata la madre dell'esproprio il ministro dell'economia Tria ha risposto che l'allora ministro Saccomanni, attuale Presidente Unicredit, subì il ricatto tedesco. L'Italia ha accettato le regole sul salvataggio interno delle banche sotto il ricatto della Germania, la quale si disse pronta a denunciare un sistema bancario prossimo al fallimento, salvo poi attenuare, dopo qualche ora, la sua constatazione già nota agli addetti ai lavori. Negli ultimi anni, signor Presidente, all'insaputa di Bankitalia e Consob, si sono verificati gli scandali di Cariferrara (con il suicidio dell'ex dirigente Paolo Bonora del 28 luglio 2015); gli allegri fidi della Banca Popolare dell'Etruria, con crediti dubbi alla clientela per 1,69 miliardi di euro; 770 milioni di sofferenze e il suicidio di Luigino D'Angelo, il pensionato che aveva perso i risparmi di un'intera vita di lavoro; per cento su prestiti, mutui e fidi che Banche Marche concedeva ad amici e compari; il commissariamento ingiusto di Carichieti e di Bene Banca, Vagienna; la Banca Popolare di Vicenza, che gonfiava il valore delle azioni fino a 62,50 euro, obbligando con metodi estorsivi a diventare azionisti; lo scandalo di Veneto Banca, che rimborsava 11.388.973 11.388.973 euro, corrispondenti a 279.482 azioni di Veneto Banca al valore di 40,75 euro euro l'una a Bruno Vespa, scavalcando 1.000 azionisti che avevano fatto richiesta prima di lui; il Monte dei Paschi di Siena, che gonfiava i bilanci con derivati Santorini ed Alexandria, spendendo 17 miliardi per acquisire Antonveneta, pagata, qualche mese prima, 6 miliardi di euro. Proprio oggi, cari colleghi, proprio oggi, ricorrono sei anni dal suicidio di David Rossi, che ha lasciato nella disperazione la moglie Antonella Tognazzi e la figlia Carolina. Sempre all'insaputa di coloro che, ben pagati, avrebbero il doveroso compito di prevenire crac e dissesti bancari, si è verificata l'incauta gestione del credito e del risparmio sanata con la risoluzione delle quattro banche. Per evitare altri crac e dissesti occorre riformare una vigilanza che non ha funzionato e che, oltre al danno, ha aggiunto la beffa di appellare i truffati quali "analfabeti funzionali" perché non sufficientemente esperti di prodotti finanziari truffaldini, proponendo l'educazione finanziaria come rimedio, alla stessa stregua di uno scippato vittima dello strappo o di un rapinato a mano armata, accusato di non avere la guardia del corpo, la licenza di porto d'armi o di non aver frequentato un corso di arti marziali. Occorre contrastare i cosiddetti intermediari vigilati per evitare di immettere sui mercati, dietro sistemi incentivanti, prodotti finanziari truffaldini e *bond* tossici piazzati agli ignari risparmiatori; evitare le porte girevoli tra vigilanti e vigilati per almeno sei anni; inasprire le norme penali per il reato di bancarotta; abrogare i premi e le buone uscite ai banchieri che hanno causato i *crac*; perseguire le responsabilità di coloro che hanno lasciato i risparmiatori in balia di se stessi. Colleghi, dalle mie parti si dice «carta canta»: ho in mano un documento, datato 30 dicembre 2015, riservato, inviato al direttorio della Banca d'Italia, che attestava che al 31 ottobre 2015, ventuno giorni prima della risoluzione delle quattro banche, su 623 miliardi di *bond*, alcune obbligazioni subordinate, quindi soggette all'esproprio - come avvenuto qualche giorno dopo

con l'arresto del vice presidente dell'Associazione bancaria italiana Berneschi, l'ex amministratore di Carige Vita, Fernando Menconi, e altri cinque dirigenti che sottraevano ingenti somme attraverso le acquisizioni di immobili e partecipazioni societarie a prezzi gonfiati, accusati e processati anche per associazione a delinquere, riciclaggio, intestazione fittizia di beni ed esportazione illecita di denaro all'estero.

(quantificati in 100 miliardi di euro, addossati alla povera gente e ai risparmiatori), con il vero e proprio dolo di Bankitalia, che, pur sapendo benissimo e da tempo dei titoli subordinati espropriabili in mano alle famiglie per il 46,1 per cento (ossia 31 miliardi di euro su 67), non ha fatto nulla per impedire la grande stangata a danno dei risparmiatori e delle famiglie. Signor Presidente, auspico che l'articolo 47 della Costituzione,

qui abbiamo una situazione più stabile, anziché quello slittamento che era un po' una sinistra metafora di quanto accadde al sistema bancario italiano dopo gli interventi di salvataggio di chi ci ha preceduto. Qui - ripeto - abbiamo una situazione più stabile. La discussione è stata molto interessante. L'ho seguita con grande partecipazione e prendendo appunti. Vorrei iniziare con una precisazione. Nella mia breve relazione non ho rilevato che non ci fosse necessità di illustrare il tema del decreto-legge Ho rilevato che mi sembrava non ci fosse un grande interesse. Mi sono permesso, da relatore (che deve essere una figura neutra), un piccolissimo accenno polemico,

la sensazione che qualche cosa di quello che ci riguarda oggi (soprattutto qualche dettaglio di quanto è stato evocato rispetto a vicende precedenti)

Voglio anche dire che scuso il fatto che spesso in Assemblea non si è attenti a chi parla, perché c'è una cosa che fuori non si sa,

noi dovremmo fare uno sforzo maggiore per spiegare ai cittadini che le leggi che si adottano in Assemblea sono il risultato di una mediazione politica lunga e complessa, che richiede tempi, che spesso sono anche quelli dell'Assemblea stessa. Cioè, se qualche collega è in giro per l'Aula a parlare con qualche altro collega, non lo fa perché manca di rispetto a me, ma lo fa perché ha necessità di raggiungere un punto di caduta su qualche cosa di cui poi magari domani ci occuperemo. Questo lo dico anche perché, laddove qualcuno ci stia osservando, è importante che sappia che noi lavoriamo e che ci sono tanti modi di lavorare. Chiusa questa premessa metodologica - mi scuso se ha rubato tempo - entro nel merito. Devo dire che, anche se alcuni colleghi hanno rilevato che la discussione generale è un momento più tecnico della dichiarazione di voto (che è ovviamente un momento più politico), questa discussione ha avuto anche dei risvolti politici. Vorrei partire da uno di questi, che ha caratterizzato le nostre opposizioni *in utroque*, cioè l'opposizione di sinistra e l'opposizione di destra. Entrambe ci hanno rimproverato di non saperci comportare bene sui tavoli europei, di non saper tutelare le alleanze, in particolare perché noi avremmo insultato i nostri alleati. Ora, vorrei fare una considerazione molto serena.

cosiddetti alleati, che onestamente non si sa bene quali siano nel quadro europeo, dal momento che noi siamo una famiglia molto composita e che, a detta di storici importanti (penso a Jones, ma se ne potrebbero citare tanti), vede proprio nella sua diversità il segno e la causa del suo relativo successo rispetto ad altre aree del Pianeta. Quindi chi siano gli alleati, non lo so. Io, come tanti altri, ho assistito negli anni passati a uno strano fenomeno meteorologico su Roma, che è una pioggia di *légions d'honneur*; e poi però assisto anche ad atteggiamenti abbastanza poco conseguenti con la nostra accondiscendenza verso i *Diktat* che provenivano dall'estero. Pensiamo adesso all'audizione del Commissario che qui è stata citata più volte, come segno della disponibilità e della maturità delle istituzioni europee, e della loro volontà di venirci incontro. Io ieri avrei voluto parlare in inglese, ma mi hanno detto che non si fa, perché siamo nel Parlamento italiano. Ma vorrei tradurre la replica della Vestager alla mia domanda.

è una cosa rischiosa, perché a suffragio universale venne salvato Barabba, allora fatalmente la mente corre a quell'episodio storico. E ieri abbiamo visto Pilato. Ieri Pilato cosa ci ha detto: "Sapete com'è andata? Purtroppo una volta il mercato delle sofferenze non c'era e quindi voi le avete cedute a prezzi stracciati mettendo in crisi il vostro sistema bancario. Adesso c'è,

che, se vogliamo veramente ragionare in termini di interesse nazionale, allora bisognerebbe fare tutti uno sforzo, ed io prometto di farlo per parte mia (in un mondo ideale dovrebbe essere così), per evitare che, quando dall'estero arrivano censure, all'interno se ne goda per usarle in modo tattico e strumentale contro la parte politica avversa. Questa cosa non funziona; è dal tempo di Carlo VIII che non funziona. Mi vedo costretto a ripetermi. Affinché certi richiami alle istituzioni europee siano credibili, dovrebbero essere affiancati da questo: che le nostre opposizioni, nel momento in cui il Paese viene insultato - e a settembre lo fu, perché si parlò di un Paese in preda a tanti piccoli Mussolini - si unissero a noi nella ferma risposta a questo tipo di atteggiamenti e non accusassero il Governo se per la prima volta reagisce. Mi rendo conto che questa è una discontinuità,

Qualcuno l'ha definita una sceneggiata, ma io con molta serenità esorterei i colleghi dell'opposizione a non valutare le nostre proposte sulla base delle loro esperienze. mi sembra che non concluse molto, e forse un motivo c'era: era una Commissione nella quale una certa parte politica giudicava sé stessa sulle politiche che aveva condotto, il giudizio della Commissione è stato positivo, quello degli elettori lo sappiamo: fine delle trasmissioni. Adesso c'è da lavorare sul serio e siccome siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è un problema di normazione, un problema di applicazione delle norme, un problema di come la vigilanza è stata esercitata - e questo tema lo vorrei affrontare più diffusamente in dichiarazione di voto - aiutateci voi a fare sì che questa Commissione di inchiesta non sia una sceneggiata, partecipando in modo costruttivo, perché nelle nostre intenzioni certamente non lo è. Sono state anche evocate e sono molto grato al senatore Grimani che lo ha fatto - la contraddizione e l'asimmetria esistenti fra una supervisione che sempre più viene portata a livello europeo come ciò è accaduto in tema bancario, perché ormai il processo è pressoché compiuto (ricordiamo che sta avvenendo anche sul tema della vigilanza dei mercati finanziari)

Come pensiamo che possa sopravvivere e possa non incrinarsi un sistema che si basa su una simile

per quel che attiene al tema generale della supervisione, noi dovremmo essere promotori in Europa di un ripensamento generale dell'approccio che viene adottato, basato sulla valutazione del rischio nella determinazione dei livelli di capitale proprio ieri sul «Financial Times» veniva seriamente messo in questione per il semplice motivo che si basa largamente su valutazioni delle banche. Siccome le banche vanno in crisi quando non sono in grado di valutare le circostanze, appoggiarsi alle loro valutazioni per decidere quale banca è in crisi comporta un dato ovvio: una rilevante sottovalutazione del rischio che poi si riflette sull'emergenza di incidenti come quelli del quale qui oggi ci dobbiamo occupare. C'è quindi proprio un problema di logica dell'approccio e questo è un problema culturale che convoca tutti noi; non è un problema di destra o di sinistra, su questo credo che saremo d'accordo. Quello che è di destra o di sinistra forse è la volontà di imporre una visione di interesse nazionale ai tavoli sovranazionali, sempre nell'ambito della solita considerazione di cornice che o l'Europa dimostra di essere un luogo efficiente per la mediazione di interessi diversi, oppure dimostra di non avere particolare ragione di esistere. risolvere con conflitti bilaterali o anche multilaterali i nostri problemi è qualcosa che in Europa abbiamo sempre fatto. Sono sempre molto scettico quando si demonizza il conflitto occorre che emerga e che sia gestito in modo efficiente. L'idea che avremo la pace per sempre ce la possiamo dimenticare. Ci saranno sempre dei problemi; il punto è

Nella mia relazione ho parlato del fatto che l'episodio del quale ci occupiamo, come tanti altri, ha due ordini di motivazioni: una motivazione di ordine generale, la recessione, della quale qui tutti oggi siamo consapevoli, e una motivazione legata alla malagestione, perché naturalmente siamo tutti umani, anche i *manager* delle banche, e possiamo essere solleciti a interessi particolari o possiamo commettere errori di valutazione. Vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea il fatto che, in uno studio di due anni fa (se non vado errato), Luigi Zingales, che è uno dei più eminenti economisti italiani,

quantitativa è la seguente: la percentuale di *non performing loan* attribuibili a fenomeni di *mala gestio* si colloca fra il 4 e l'8 per cento.

E allora, se il problema è sistemico, questo esalta la considerazione fatta dal collega Grimani, perché i problemi sistemici, che in un mercato finanziario interrelato e integrato come quello che abbiamo voluto costruire (forse con una certa avventatezza) qui in Europa necessariamente dipendono anche dai comportamenti di operatori in altri Paesi, non possono essere lasciati, quando si tratta di risolverli, unicamente sulle spalle delle autorità e delle collettività nazionali.

Questo è un tema politico, a mio avviso, anche se ci sono dei dati di fatto che vanno messi in evidenza per verificare se veramente questo episodio sia la fotocopia di altri episodi. Magari di questo preferirei parlare con maggiore ampiezza in fase di dichiarazione di voto. Qui vorrei sollevare, avviandomi a concludere, un altro tema di carattere che ho visto emergere in moltissimi interventi nel corso della discussione generale (non cito i colleghi, perché ritengo che sia meglio non farlo). al tema della tutela del credito locale. Ognuno di noi ha esperienze nei propri collegi e sa cosa significa quando le istituzioni del credito territoriale incorrono in situazioni di crisi. Sa cosa significa questo per il mondo della piccola e media impresa e sa cosa significa questo per gli artigiani e per le famiglie

Io non capisco molto quando viene detto che dobbiamo affidarci al mercato più che alle banche e che dobbiamo sostituire il debito con il finanziamento sul mercato. Certo, la parola debito ha una valorizzazione negativa e quindi è chiaro che, nel momento in cui il credito bancario viene chiamato debito, già lì è implicito che si vuole mettere l'interlocutore in una posizione di inferiorità tattica e che si vuole demonizzare il lavoro che gli istituti di credito fanno in quanto intermediari bancari. Ma ci vogliamo ricordare del fatto che il mercato, quello su cui strutturalmente si finanziano le grandi aziende, sbaglia e sbaglia pesantemente? Sbagliano le banche, ma anche il mercato, che spesso sbaglia di più. La crisi di Wall Street o della Lehman Brothers sono state crisi di mercato e hanno lasciato cicatrici profonde sulla storia economico-finanziaria mondiale.

e finanziatore delle buone pratiche aziendali perché non è così nei fatti e non è così neanche nella volontà - forse dovrei dire - nella capacità operativa del regolatore europeo, che ieri è venuto qui a dirci che lui non si preoccupava del fatto che, per esempio, la gestione delle sofferenze fosse in mano a un oligopolio. L'oligopolio non è il mercato, ma un posto dove quattro o cinque persone si mettono d'accordo per fare il prezzo. Mi avvio a concludere. Credo di aver risposto a pressoché tutti i temi sollevati. Torno, però, sull'esigenza di tutelare il credito territoriale, il patrimonio delle casse di risparmio e il patrimonio delle banche di credito cooperativo, è fortemente avvertita da questo Governo, tanto più in un momento in cui vediamo profilarsi all'orizzonte un nuovo rallentamento dell'economia mondiale e in cui è assolutamente indispensabile che la parte sana della nostra economia reale non sia affidata all'isteria collettiva dei cosiddetti mercati, ma sostenuta da un sistema creditizio vicino ai territori e alle loro esigenze. *(Applausi

Signor Presidente, proverò a rispondere a qualche affermazione che ho sentito durante la discussione qui in Senato.

ho preso un po' di appunti perché neanche ricordavo queste cifre così importanti - 870 milioni, più 1,7 miliardi dati al Fondo di solidarietà. Nel decreto per le quattro banche gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati hanno visto azzerati i loro risparmi. Questo decreto non prevede un azzeramento dei risparmi per nessuno e questa è la prima differenza.

Stessa cosa sulle banche venete, dove l'azzeramento è stato di 2,5 miliardi: i capitali messi a disposizione del Fondo Atlante sono stati di 2,5 miliardi e successivamente di 938 milioni. Ricordiamo che Cassa depositi e prestiti è un'azienda partecipata dal pubblico, anch'essa ha partecipato a Fondo Atlante e ha perso tutti i soldi,

Noi cittadini italiani abbiamo dovuto regalare a questa banca ben 4,8 miliardi di euro e successivamente abbiamo dovuto mettere oltre 6 miliardi di euro a garanzia: ben 11 miliardi di soldi pubblici messi a disposizione per il sistema bancario,

Un'altra differenza importante è che su MPS non potevate fare più nulla, perché siete arrivati troppo tardi. E la forza e la bravura di questo Governo sono quelle di arrivare prima

senza arrivare al limite della ricapitalizzazione precauzionale. Se fossimo arrivati tardi, come in precedenza, saremmo stati costretti a mettere in piedi immediatamente una ricapitalizzazione precauzionale con soldi pubblici. Quindi anche che siamo arrivati prima, rispetto ad altri interventi sul sistema bancario degli ultimi cinque anni, è storia.

sul decreto un po' di attacchi da parte di alcuni esponenti politici del mio Gruppo parlamentare, ma non vi è ingerenza all'interno dell'attività

a marzo 2018 e siamo al Governo dal giugno 2018; se qualcuno avesse dovuto fare un intervento, avrebbe dovuto farlo negli anni precedenti, visto che Carige da anni metteva in piedi aumenti di capitale e continuamente ne necessitava di nuovi. Quello che abbiamo fatto noi, appena arrivati al Governo, è stato mettere una lente d'ingrandimento su questa banca;

che hanno permesso che quella banca non fosse dichiarata insolvente. Allora sì che abbiamo potuto mettere in piedi questa garanzia sull'emissione obbligazionaria,

ritirato tutti gli emendamenti. Questo quindi è il motivo: non una contrarietà nel merito degli emendamenti, ma un metodo che anche voi ci avete chiesto di mettere in piedi. Per questo motivo, la maggior parte degli ordini del giorno che ho visto, che sono assolutamente in linea con le idee del Governo, verrà

la Presidenza, in conformità con quanto stabilito durante l'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 7.4, 11.0.1, 14.3, 21-*bis*.0.2 e 21-*bis*.0.6 per estraneità all'oggetto del decreto-legge. Ai sensi della medesima norma regolamentare, risultano altresì improponibili gli emendamenti 22.0.100, 22.0.101 e 22.0.102, 22.0.102, presentati solo in Assemblea e diretti a modificare il Testo unico bancario in materia di gruppo bancario cooperativo.

luce di tutte le barzellette che ci sono state raccontate su quanto sono bravi e belli e di tutti i riferimenti sciocchi e fuori luogo che sono stati fatti in quest'Aula, mi domando e le chiedo formalmente: siamo tranquilli su questo provvedimento? È confermata

di organizzare immediatamente una riunione della Conferenza dei Capigruppo, dato che a differenza di questo Governo e di questa maggioranza, noi abbiamo a cuore il futuro

Senatore Marcucci, allo stato attuale non ho alcuna novità sulla tempistica. Siamo arrivati all'illustrazione degli emendamenti e per quello che mi riguarda, durante il mio turno di Presidenza, proseguiamo con tale illustrazione.

Grazie, che secondo lei, Presidente, l'emendamento 7.4 è estraneo alla materia. Mi domando per quale motivo sia estraneo alla materia un emendamento che dovrebbe stare a cuore a moltissimi senatori presenti in Aula o o rappresentanti della maggioranza, che chiede semplicemente di introdurre delle norme di carattere etico per gli stipendi e le remunerazioni dei dirigenti delle banche salvate dallo Stato. Noi abbiamo assistito non soltanto allo scandalo della mancata vigilanza da parte di Banca d'Italia

si prende l'impegno di salvare le banche e di mettere a disposizione garanzie pubbliche, che sono pagate con i soldi dei cittadini, degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti, perché allora è estraneo allora è estraneo alla materia il principio per cui i nuovi amministratori devono avere compensi non superiori al massimo del compenso attribuibile ad un alto dirigente dello Stato? che dopo aver salvato le banche e i risparmiatori si torni alla prassi scandalosa di amministratori incapaci e forse anche disonesti che percepiscono 2, 3, 4, 5 milioni di euro all'anno, mentre un dipendente della banca, sì e no, arriva a 2.000 euro

stata dichiarata in Commissione e lei ne aveva conoscenza.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la seduta riprende con la discussione delle mozioni all'ordine del giorno. Seguiranno le dichiarazioni di voto e la votazione finale sul decreto-legge concernente la Banca Carige, anche oltre l'orario di chiusura della seduta stabilita da calendario.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi ci troviamo a discutere della mozione di cui sono primo firmatario ed a cui hanno aderito tantissimi colleghi di diversi Gruppi parlamentari;

mi preoccupa, perché oggi rischiamo di prendere una decisione facendo prevalere gli interessi dei partiti, invece di quello del Paese e degli oltre 70 milioni di persone di origine italiana che vivono nel mondo. Il Comitato è stato istituito nel corso delle passate legislature, dalla XIV alla XVII, al Senato e alla Camera dei deputati, con il compito di approfondire condizioni, problemi e aspettative delle collettività italiane residenti all'estero. Alla Camera dei deputati il Comitato è stato recentemente istituito anche per la XVIII legislatura. Non capisco come possiamo non fare lo stesso anche al Senato della Repubblica. Il ruolo rivestito dal Comitato in questi anni è stato di fondamentale importanza sia per il Parlamento che per le nostre comunità all'estero. Sono stati acquisiti elementi conoscitivi su problematiche ed aspettative, valutando come contribuire alla loro soluzione con interventi normativi e contatti con istituzioni italiane ed autorità straniere. Tra i tanti temi esaminati ricordiamo la valorizzazione del contributo economico, culturale e civile delle comunità italiane all'estero, servizi consolari, promozione della lingua e cultura, riforma della legge sulla cittadinanza ed analisi di questioni specifiche come gli effetti della Brexit sulle comunità e sull'Italia. Penso che nessuno di questi temi sia prerogativa di un singolo partito o di una parte del Parlamento. L'elezione dei parlamentari nella circoscrizione Estero ha consentito al Parlamento la possibilità di creare un nuovo rapporto con le comunità italiane nel mondo. In maniera autocritica, però, credo che in questi anni non siamo purtroppo riusciti - mi riferisco agli eletti all'estero - a far capire al Parlamento e al Paese tutto il grande potenziale di una collaborazione attiva con le nostre comunità nel mondo. Il settore portante dell'economia italiana è l'*export* del *made in Italy*. Nessuno può mettere in dubbio il ruolo degli italiani nel mondo per aver contribuito a definire lo stile di vita delle comunità ospitanti, facilitando così l'ingresso di beni e servizi italiani. In altre parole sono stati gli ambasciatori non pagati del sistema Paese. Oggi le nostre comunità sono mature ed integrate in moltissime delle società ospitanti; i nostri figli e nipoti ricoprono ruoli ed incarichi importanti in tutti i settori della società. Immaginate la differenza tra operare in mercati dove vi sono persone orgogliose delle proprie origini italiane o cercare di entrare in nuovi mercati dove lingua e cultura italiana sono conosciuti solo tramite libri di testo? Ecco, chiedetelo ai rappresentanti delle tantissime imprese italiane coinvolte in processi di internazionalizzazione perché loro sanno qual è la differenza. Dentro le istituzioni italiane molto spesso non ce ne rendiamo conto, malgrado la presenza dei parlamentari eletti all'estero. Certamente iniziative come l'indagine conoscitiva sulle condizioni e le esigenze delle comunità degli italiani all'estero, recentemente autorizzata alla Commissione affari esteri, emigrazione, costituiscono un valore aggiunto ai lavori del Senato, ma questa da sola non basta e non si può sostituire al Comitato. Si tratta di un'iniziativa specifica che non permette di avere una visione globale e continua sui tanti temi d'interesse e sulle potenzialità delle nostre comunità all'estero per la promozione del sistema Paese. Occorrono scambi di opinioni, idee e metodologie di lavoro per tutta la durata della legislatura, cosa che solo il Comitato è in grado di fare. Tanti sono i temi di attualità sul tappeto, che rischiano di non essere approfonditi e ai quali, senza un organo istituzionale specifico, rischiamo di dare delle risposte legate all'iniziativa personale di chi nel momento si sente più coinvolto, oppure di chi crede di ottenere vantaggi politici. Temi che assumono aspetti diversi, a volte opposti, a seconda delle aree geografiche dove i nostri connazionali si sono stabiliti e continuano a stabilirsi. Tra questi ricordo l'assistenza ai connazionali che vivono nei Paesi in crisi, l'attuazione e la revisione di accordi previdenziali e di assistenza sanitaria, servizi consolari, assistenza alle nuove migrazioni, gli effetti della Brexit, il riconoscimento all'estero di titoli di studio, ed in particolare le qualifiche professionali italiane, la copertura previdenziale per gli italiani che nel mondo globalizzato si muovono da un Paese a un altro, specie in Paesi asiatici, africani e dell'Oceania, dove non esistono sistemi pensionistici di tipo previdenziale. Ci sono poi i temi della promozione del sistema Paese. Nella mia vita accademica e professionale ho imparato che il singolo fattore che contribuisce più di tutti al successo dei processi di internazionalizzazione è la fiducia. La fiducia non è una cosa che può essere imposta, ma va guadagnata sul campo imparando a conoscersi a vicenda. Nelle relazioni internazionali la base per conoscersi è capire e rispettare le differenze culturali. Lingua e cultura sono il primo passo per capirci meglio: promuovere l'insegnamento della lingua italiana nel mondo ed organizzare iniziative culturali atte ad avere un impatto nelle società locali sono temi fondamentali. Come ripeto *ad nauseam*, si tratta di un investimento nel futuro, non di spesa corrente. Il grandissimo *network* degli italiani nel mondo, di cui parlavo prima, costituito dai nostri figli e nipoti, che ricoprono ruoli decisionali importanti nelle società ospitanti, può essere un'altra grande risorsa. infatti facilitare l'ingresso del *made in Italy* nei loro Paesi di residenza e l'espansione nei Paesi limitrofi o possono permettere di individuare temi per stabilire una più stretta collaborazione tra l'Italia e i loro Paesi: sto pensando, per esempio, agli effetti della Brexit sui Paesi dell'Oceania. Signor Presidente, potrei

Anche alla luce dell'importante ruolo svolto dal Comitato nelle passate legislature, l'istituzione nella XVIII legislatura al Senato è a mio avviso un dovere nei confronti dei nostri connazionali all'estero e un servizio alla società italiana. di una scelta politica che fa da spartiacque fra chi ha interesse e ha a cuore gli italiani nel mondo e chi, da un lato, predica interesse ma, dall'altro, pratica indifferenza. Oggi, con l'approvazione della mozione in esame, abbiamo la possibilità di continuare a mantenere vivo il collegamento con i nostri connazionali all'estero. Abbiamo la possibilità di mandare un segnale forte, di un impegno da parte del Parlamento e delle istituzioni italiane nei loro confronti, di ribadire la consapevolezza che essi sono per l'Italia una risorsa economica, sociale, culturale e politica. Signor Presidente, concludo auspicando la più ampia convergenza da parte dell'Assemblea sulla costituzione del Comitato.

una questione immediata, che a mio avviso richiede una certa attenzione. Sto parlando dell'esercizio di voto della comunità degli italiani nel Regno

Grazie, signor Presidente. per sollevare una questione più urgente e immediata, riguardante la comunità italiana nel Regno Unito e l'esercizio di voto per le elezioni

Nell'incertezza totale su quello che può succedere (Brexit sì o Brexit no, *deal* o *no deal*), è chiaro che questi nostri connazionali si sono già rivolti al Governo con una lettera pubblica

ha dato piena disponibilità e ha dichiarato di essere operativamente pronta a far loro esercitare il diritto di voto nel Regno Unito. Il ministro Salvini, rispondendo all'interrogazione di cui le dicevo, ha dichiarato che la competenza è del Ministro degli affari però per quanto di sua competenza (del ministro Salvini) ha risposto dando la massima disponibilità e apertura anche a rivedere eventuali normative, vista l'eccezionalità della situazione. Vorrei richiamare l'attenzione proprio sulla eccezionalità della situazione,

Insisto quindi a dire che anche un intervento temporaneo e parziale di adeguamento della legge n. 408 del 1994, vista la straordinarietà della situazione, a mio avviso non solo consente ma implica anche un intervento straordinario per dare ai nostri cittadini almeno qualche certezza su come si devono comportare. nel confermare il voto favorevole all'istituzione del Comitato, ci terrei a segnalare un problema urgentissimo, perché mancano poche settimane. Vedo la disponibilità del Ministro dell'interno;

Grazie, Presidente.

del Paese sparse per il mondo, persone che vivono nel loro DNA l'essere proiettate verso orizzonti internazionali e che vivono la globalizzazione nel loro quotidiano. Tra l'altro, parliamo di concittadini spesso perfettamente integrati nei luoghi di residenza; a volte sono addirittura eccellenze nei vari ambiti dell'imprenditoria, del sapere, della ricerca, della cucina, dell'enogastronomia e dell'*import-export*.

essi sono profondamente radicati alle loro radici italiane: dunque, una grande potenzialità per il sistema Paese nel mondo. Un fenomeno che, proprio negli ultimi anni, ha conosciuto numeri estremamente importanti, per tanti versi addirittura equiparabili a quelle che furono le ondate migratorie più consistenti del nostro Paese negli anni Sessanta-Settanta, del *boom* economico. Tra l'altro, un fenomeno che non riguarda soltanto i singoli destini personali di questi nostri concittadini che hanno ripreso massicciamente ad andare all'estero, ma che è sempre più un fenomeno che riguarda il Paese, che interessa anche i luoghi di partenza,

rappresenta anche un costo per il Paese. Se, infatti, in passato, fino agli anni 2000, la maggior parte di coloro che partivano erano persone con bassi titoli di studio (pensate che, fino al 2000, cento di chi andava all'estero era dotato, al massimo, di un titolo di licenza media), oggi i dati sono di altro tenore. Oggi, ben un terzo dei connazionali che partono sono laureati o, addirittura, dotati di titoli di studio ancora più elevati, come, ad esempio, dottorati allora, il Comitato degli italiani nel mondo anche qui al Senato? Perché questo fenomeno interessa in misura particolare proprio il Paese,

dell'impatto della legislazione in materia di italiani all'estero. Un esempio fra tutti: proprio stamane giornali nazionali riportano, in merito a una proposta di legge adottata dal Parlamento una decina di anni fa, tra l'altro in modo *bipartisan*, la famosa legge Controesodo,

c'è bisogno, anche a livello legislativo, all'interno dell'istituzione del Senato, di un organo istituzionale *ad hoc*, finalizzato espressamente a valutare, anche dal punto di vista normativo, quali provvedimenti possano essere messi in campo

accanto a tutti quelli già enunciati dal collega Giacobbe, rispetto a potenziali ambiti di cui il Comitato per gli italiani all'estero potrebbe e dovrebbe rendersi interlocutore. Un altro esempio potrebbe essere favorire il reinserimento di tanti nostri medici specialisti operanti all'estero per far fronte a quella forte difficoltà che stanno conoscendo le nostre strutture pubbliche di carattere sanitario, proprio rispetto a numeri allarmanti di *deficit* e carenza

ben 10.000 medici specializzati formati dalle nostre università, tra l'altro con costi consistenti. Basti pensare che

che poi, magari, una volta formato, si è recato all'estero. Negli ultimi dieci anni contiamo ben 10.000 giovani risorse che si sono trasferite all'estero per esercitare la professione di medico specialista,

addirittura senza accordo, quindi con un *no deal*, si rischia, all'indomani del 29 marzo, di vedere tantissimi nostri giovani cervelli, oggi perfettamente inseriti nel contesto locale, essere privati del loro *status* *status* giuridico di cittadini europei. Signor Presidente, questo era soltanto un esempio - anche molto concreto - per ribadire quanto un organo istituzionale come il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, istituito qui al Senato,

un lavoro di proposta politica e legislativa nei confronti del Parlamento italiano. Mi auguro, dunque, signor Presidente, che ci siano ancora gli elementi politici affinché il Governo prenda seriamente in considerazione l'ipotesi di costituire questo Comitato. Ci auguriamo che il fatto che siano state ritirate le firme dalla sottoscrizione della mozione da parte del MoVimento 5 Stelle non non preannunci un potenziale atteggiamento ostile del Governo perché questo, come diceva benissimo il collega Giacobbe, sarebbe il segnale di una disattenzione non tanto nei confronti del Partito Democratico, promotore della mozione, bensì di tutte le nostre comunità di italiani all'estero, le quali auspicano, invece, che ci possa essere un lavoro bipartisan, che si renda conto di quanto le nostre comunità siano un grande valore, *in primis* per il Paese. *(Applausi

Signor Presidente, il Governo ovviamente attribuisce la massima attenzione alle comunità italiane all'estero, che rappresentano una risorsa economica, sociale, culturale e politica del nostro Paese. Le politiche a favore degli italiano all'estero, compresi coloro soltanto temporaneamente residenti all'estero, costituiscono un aspetto fondamentale della politica estera italiana. Si tratta di un tema al quale in particolare Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attribuisce una centralità strategica, e che vede impegnati i nostri uffici centrali e la nostra rete diplomatico-consolare per fornire servizi consolari, assistenza ai connazionali e nel promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiane. italiane. Vorrei assicurare e garantire a tutti che il Governo, a prescindere dalla dinamica parlamentare che oggi sarà in quest'Assemblea, attribuisce la massima attenzione al tema, e lo farà in un caso o nell'altro. Il segnale di attenzione, d'altronde, è stato già dato anche nell'ultima manovra economica, attraverso la quale, per la prima volta dopo tanti anni, si è riusciti ad assumere al Ministro degli affari esteri 350 persone, tra cui 50 contrattisti destinati proprio alle sedi estere per poter fronteggiare fenomeni come la Brexit e la richiesta costante di maggiori risorse per consolati come quelli dell'area latinoamericana, ad esempio. Soprattutto, si è riusciti a inserire un aumento della dotazione economica riferita ai contrattisti per permettere ai nostri Consolati di avere personale che lavora a pieno regime laddove c'è davvero bisogno.

per fornire a tutti gli italiani all'estero un percorso da seguire qualunque sia lo scenario. Aggiungo che, sempre nell'ultima manovra, è stato ribadito l'impegno per il piano promozionale a favore dell'Italia, che non è soltanto economico, ma anche relativo alla promozione

ci siamo già portati avanti per garantire il voto consolare nel caso in cui ci sia una richiesta di prolungamento *ex* articolo 50 (quindi, sostanzialmente, qualora ci sia ancora questa fase di stagnazione).

in difficoltà nel credere a quello che, dal nostro punto di vista, doveva essere buono e giusto per tutti. Quando la mozione fu presentata, ci sembrava la cosa più naturale del mondo. Dico questo anche al rappresentante del Governo, che prima ha spiegato alcune questioni,

attivamente - lo dico e vorrei che il Governo ne prendesse atto - anche per rendere efficaci quelle misure di cui oggi il sottosegretario Merlo, che mi spiace non vedere in Aula,

agevolare misure che il Governo aveva adottato nei confronti degli italiani all'estero, in modo particolare per la diffusione della lingua italiana. Ricordo la legge delega n. 107 del 2015, che garantiva uno spazio d'azione molto particolare, ma dall'altra parte ricordo anche quegli emendamenti sottoscritti con forza dagli eletti all'estero, e non solo, che avevano portato alla ripartizione di un fondo, quello di cui oggi - lo ripeto - il sottosegretario Merlo si prende i meriti, che garantiva 50 milioni ogni anno proprio per questo tipo di

noi non abbiamo avuto segnali da parte di questo Governo, se non belle parole nei confronti degli italiani all'estero. Ma segnali concreti non ne abbiamo. Glielo dico perché di parole siamo anche un po' stanchi, anche un po' stanchi, e siamo stanchi - glielo ribadisco - perché nella misura in cui lei prende con grande facilità l'impegno con la senatrice Bonino rispetto alla questione dei nostri connazionali, che vivono una situazione molto particolare per quanto riguarda la Brexit, e quindi nel Regno Unito, le sue parole non sono per nulla di tranquillità e di garanzia. Vorremmo qualcosa in più, perché il piano B forse voi dovreste incominciare a preannunciarlo e non semplicemente dire che sareste quasi disposti a togliere un diritto, ossia di poter votare lì dove sono, lavandovene tranquillamente le mani perché vi risulta il modo più semplice. Abbiamo avuto quattro legislature con questo

Solo che noi ci siamo resi conto che questo Governo non ha fatto altro che spartirsi in maniera equa posti e poltrone. Non vorremmo che in questa circostanza si sia spartito anche le Camere, e quindi, poiché la Camera ha

Purtroppo non riusciamo a pensarla in maniera positiva nei vostri riguardi; la vostra miopia non vi fa vedere nei confronti degli italiani all'estero quell'opportunità che invece noi riteniamo essi siano e di cui siano portatori. Non vi sentiamo mai parlare, infatti, della grande opportunità che gli italiani all'estero possono dare al sistema Paese Italia, grazie alla loro capacità di creare *network* e di creare rete. I nostri imprenditori hanno bisogno anche di quella base all'estero, che dal vostro punto di vista non merita assolutamente di essere valorizzata. Forse perché voi avete in mente una figura degli italiani all'estero molto diversa da quella che, ad esempio, la collega Garavini e il collega Giacobbe vi hanno illustrato prima, ossia di un mondo estremamente complesso ma con molte risorse, pronto a mettersi in gioco per il proprio Paese di provenienza (se il proprio Paese di provenienza avesse il buon gusto di

rende incapaci di vedere e leggere le problematiche che i nostri connazionali stanno vivendo. Lo dico con la consapevolezza di chi è stata italiana all'estero, perché ho vissuto in Germania e anche in Croazia e ho avuto l'opportunità di vedere qual è il ruolo che le comunità italiane svolgono nel fare ponte, nella possibilità di trovare contatti, anche nel semplice modo di facilitare le questioni burocratiche. Un Comitato come quello che potrebbe nascere al Senato serve anche per migliorare questo sistema, perché ha proprio la funzione di portare avanti dei progetti che siano veramente *ad hoc*, che diano l'opportunità di parlare di quel tema, che risolvano il problema nella sua specificità, altrimenti passa sempre tutto in secondo piano, diventa uno dei tanti commi che si trovano all'interno della legge di bilancio, diventa uno dei tanti emendamenti senza progettualità, senza costruzione, proprio secondo quella regola di improvvisazione che invece vi caratterizza. C'è un altro aspetto che mi preoccupa

che la possibilità di questo Comitato di fare anche indagini di natura conoscitiva, di valorizzare le belle esperienze delle nostre comunità all'estero che portano con sé delle storie grandi di integrazione, integrazione, turbasse gli animi di qualche collega che invece pensa che l'integrazione non sia una ricchezza e che invece vive sempre il principio di mescolanza non tanto come un'opportunità, ma come un pericolo. Con questa moda del sovranismo, del guardare sempre e solo in casa propria, nella visione di un'italietta ristretta all'interno dei propri confini, tutto ciò che arriva dall'esterno diventa pericoloso, e allora guai,

più numerosa al mondo - che queste buone pratiche e questi buoni esempi potessero far cambiare idea a qualcuno. Temo che in questa vostra miopia ci sia anche l'assoluta mancanza di coraggio di dire che alcune volte conoscere e farsi portatori di un patrimonio di esperienze, che magari molti all'interno di quest'Aula non conoscono, sia una ricchezza e non una paura da combattere. *(Applausi

sostanzialmente non tiene minimamente in conto l'importanza e gli interessi degli italiani attualmente residenti all'estero. Questa cosa io la voglio smentire, perché a dispetto di chi parla di miopia su questo argomento, voglio ricordare - e lo ricordo a me stesso, che ho parte della mia famiglia che è residente all'estero che vive quella situazione in prima persona, esattamente dall'altra parte del mondo - che so esattamente cosa vuol dire far parte di una comunità importante,

Parliamo di un'altra cosa, parliamo di un organo che dovrebbe preoccuparsi di seguire queste problematiche, ma abbiamo appena sentito proprio dal Sottosegretario che queste problematiche vengono seguite e c'è un impegno formale in questa sede (ricordiamoci che siamo al Senato). E ha appena detto che la problematica degli italiani all'estero non è una problematica di secondo piano. Questo secondo me è molto importante; però molti probabilmente non lo vogliono sentire, ma vogliono semplicemente buttarla in polemica, là ove non c'è proprio nulla.

Abbiamo recentemente approvato un'indagine conoscitiva in Commissione plenaria; ciò vuol dire che la Commissione affari esteri, emigrazione si occuperà di queste problematiche.

Ebbene, evidentemente, se il fenomeno si è accresciuto in questo modo, bisogna anche modificare gli strumenti con cui andiamo ad approcciare questo problema. Noi riteniamo che l'indagine conoscitiva che abbiamo recentemente approvato in Commissione, e che è stata approvata dalla Presidenza del Senato, sia uno strumento

Alla Camera, come giustamente è stato ricordato, c'è un Comitato. Benissimo. Al Senato, vogliamo provare a capire se lo strumento che precedentemente era corretto lo è ancora? Probabilmente oggi non lo è più, perché è cambiato il fenomeno. E questo non vuol dire tenere in secondo piano gli interessi degli italiani all'estero. Io continuo a sentire questo argomento, che ritengo profondamente ingiusto, perché abbiamo comunque dei Gruppi parlamentari che si sono impegnati nelle apposite sedi per tenere in debito conto questa situazione.

non meriti polemiche, ma meriti essenzialmente degli interventi concreti, quegli interventi che venivano auspicati e sui quali sono d'accordo: mantenere il collegamento, mantenere mantenere proficuità rispetto a questo rapporto. Sull'*import-export* e sui rapporti economici sono assolutamente d'accordo; sono costantemente in contatto con molte realtà e sottoscrivo questa cosa. Ma non credo che mettere sullo stesso piano problematiche degli italiani all'estero e l'istituzione di un Comitato sia una questione così dirimente, proprio perché l'impegno del Governo e l'impegno del Parlamento rimangono fermi su questa problematica e sulla situazione degli italiani all'estero. Credo che questo sia fondamentale. l'interesse del Paese, poc'anzi si ricordava che è interesse del Paese la costituzione di un Comitato (riassumo, ovviamente). Io credo che l'interesse del Paese sia mantenere una propria identità mantenere il collegamento con coloro che vogliono mantenere un legame con il proprio Paese natio. Il Comitato sarebbe semplicemente uno strumento, ma, come dicevo prima, probabilmente è ora di cambiare ed è ora di sperimentare altri strumenti. Non accetto nemmeno - lo dico nel totale rispetto delle posizioni avverse - che questo venga considerato come uno spartiacque tra chi ha interesse a tutelare a tutelare gli italiani all'estero e chi invece non gliene frega niente. Io questo non lo non lo ritengo corretto, non lo ritengo accettabile e non lo condivido. È per questo - non voglio dilungarmi oltre - che

anzi, è uno sprone per noi, perché vuol dire coinvolgere tutta la Commissione affari esteri, emigrazione a lavorare meglio e più alacremente e a mantenere contatti più profondi, che altrimenti rischierebbero di rimanere relegati solo a un comitato. Invece noi vogliamo andare oltre. Io invito chi non è d'accordo con noi su questo aspetto a leggere la questione da questo punto di vista, perché questo è l'unico punto di vista che ci pone alla base del fatto che noi non riteniamo attualmente di sostenere la costituzione del Comitato.

che, tra l'altro, confonde il piano del Governo con quello del Parlamento. Non sono stupito del fatto che a rappresentare la posizione del Governo

varie esperienze e condivide questa causa. Come dicevo, però, non sono stupito del fatto che ad esprimere la posizione del Governo non favorevole alla ricostituzione del Comitato per le

Ricordo che siamo in un sistema bicamerale e che la Camera dei deputati ha istituito per l'attuale legislatura, come per le quattro precedenti, il Comitato per gli italiani nel mondo.

abolire di fatto l'unico Comitato dedicato specificamente alle questioni degli italiani all'estero; non ci sono altre storie. L'indagine conoscitiva citata dalla Commissione affari esteri è uno specchietto per le allodole che ha dei caratteri istituzionalmente scandalosi. Non si fa un'indagine conoscitiva sul 10 per cento della popolazione italiana: si fa un'indagine conoscitiva sui fatti del Forteto o comunque su qualcosa di estremamente circoscritto, ma non sugli italiani all'estero e voi lo sapete tutti, perché tutti avete qualche collegamento con qualcuno residente all'estero. Gli italiani all'estero sono il 10 per cento della popolazione e, che lo vogliate o no, meritano rispetto, meritano un Comitato che abbia come *focus* l'analisi e la promozione delle nostre tematiche.

un'azione *bipartisan* diretta dal centrodestra, dal ministro Tremaglia (che si starà rivoltando nella tomba), ha consentito che si desse un rilievo istituzionale ad un fenomeno come quello migratorio italiano che non ha eguali nel mondo. Gli italiani sono emigrati per due secoli e continuano a farlo: ogni anno ne spariscono 150.000. Pensate ai vostri territori e immaginateli con 150.000 persone in meno il prossimo anno.

faremo il conto di quanto sono stati utili agli italiani all'estero. Con lo stesso criterio potete assumere 50 nuovi ambasciatori e dire che lo fate per gli italiani all'estero. Al momento sono solo parole. Dopodiché sia chiaro: quattro legislature. Non approvando questo Comitato, fareste come quei talebani che, siccome hanno il controllo del territorio per un certo periodo, fanno saltare tutti i monumenti e le opere d'arte realizzati da civiltà precedenti. Avete il controllo del Parlamento in questo momento? Benissimo; lo utilizzate per far fuori

l'abolizione del Comitato per gli italiani all'estero. Non ho visto nel nostro programma la riduzione dei rappresentanti della circoscrizione estero. Sono andato a controllare e non c'era questo punto neanche nel programma dei 5 Stelle, che pure è stato premiato della fiducia di 150.000 elettori. Avete chiesto e ottenuto la fiducia di 150.000 italiani residenti all'estero sulla base di un programma che non diceva che avreste abolito il Comitato per gli italiani all'estero. Non diceva che avreste ridotto la rappresentanza parlamentare addirittura a quattro senatori per 6 milioni di persone. Vi segnalo peraltro che gli italiani all'estero non sono quelle macchiette che continuate a dipingere, specie i *media* di questo Paese. Sulla questione della riforma costituzionale riduzione del numero dei parlamentari proporremo un'eccezione alla Corte costituzionale. Non aspetteremo che la Corte costituzionale invalidi la legge *ex post*, ma proporremo un ricorso. Il giudice Cartabia nell'ordinanza n. 17 del 2019 ha dato questa possibilità e noi intendiamo sfruttarla fino in fondo. Bloccheremo questo disegno di legge nefasto e non vi permetteremo, finché saremo qui, di vietare agli italiani all'estero l'esercizio dei propri diritti politici. Concludo raccomandandomi al fatto che siete tutti parlamentari della Repubblica, siete tutti senatori: questa è una decisione del Senato della Repubblica che produrrà

eletto di cui questo Paese deve andare fiero. Loro saranno i megafoni della decisione che state per prendere: quindi abbiate rispetto e considerazione per questa materia e per gli italiani residenti all'estero, perché non è solo per il fatto che adesso controllate questo Parlamento che potete rinnegare i loro diritti.

Signor Presidente, il senatore Fantetti che mi ha preceduto ha detto praticamente tutto ciò che c'era da dire su questa materia e Fratelli d'Italia si associa pienamente alla sua dichiarazione. Vorrei

Chi è vissuto all'estero e ha fatto una qualunque esperienza all'estero o chi ha un'attività commerciale che si relaziona con l'estero sa bene che la presenza delle comunità italiane all'estero sono una enorme ricchezza politica e commerciale per l'Italia. Tutte le Nazioni investono cifre ingenti per creare un tessuto di rapporti commerciali e politici d'interesse nei diversi Paesi del mondo,

L'Italia da sempre utilizza le proprie comunità all'estero come contatto diretto nei diversi Paesi del mondo. Un imprenditore che voglia investire in Argentina avrà un'enorme facilità, perché lì troverà associazioni

non ci vuole proprio un genio per capire che le nostre comunità all'estero sono per noi una ricchezza. La faccenda di aver riconosciuto il diritto di voto agli italiani all'estero certo

*forma mentis* sostiene che la Nazione italiana non sia limitata a chi ha la cittadinanza italiana, ma sia un concetto più ampio; c'è però anche un risvolto di utilità e di ritorno di ricchezza per l'Italia, che è quello che dicevo prima.

dovrebbero rafforzare l'enorme particolarità dell'Italia, ossia le proprie comunità all'estero. Sempre chi ha avuto a che fare con i rapporti con l'estero sa, ad esempio, quanto ogni singola Nazione europea spenda per aprire scuole in giro per il mondo. Infatti, chi

nella cui cultura si è formato negli anni della scuola, cosa che diventa una ricchezza a tempo indefinito per chi ha aperto quelle scuole.

Concludo dicendo semplicemente che rinunciare ai rapporti con le nostre comunità all'estero è un atto grave che continua a indebolire l'Italia nei nostri confini e all'estero. Per questo motivo, Fratelli d'Italia voterà ovviamente a favore della mozione per la costituzione del Comitato per gli italiani all'estero.

il mio intervento, che illustrerà le ragioni del no a questa mozione, presentata dal senatore Giacobbe e da altri senatori, s'incentra su due parole chiave, la prima delle quali è inesattezza e la seconda è autoreferenzialità. Cominciamo dalle inesattezze, perché ne sono state dette diverse in quest'Aula, a partire soprattutto da una: agli italiani residenti all'estero certo non interessa che qui al Senato si dia l'avvio a un Comitato, con l'istituzione di nuove poltrone. Agli italiani residenti all'estero interessa che funzionino i servizi per le nostre comunità. L'altra inesattezza ripetuta più e più volte, non soltanto oggi, ma anche in Commissione affari esteri, emigrazione, riguarda la formazione del Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema Paese alla Camera dei deputati. come si può vedere aprendo il sito, non si tratta di un Comitato autonomo, ma si tratta di un sottocomitato della Commissione affari esteri della Camera, composto da 21 deputati tutti della Commissione affari esteri. Arrivo all'altra questione che riguarda l'istituzione del Comitato. Signor Presidente, anch'io, come il senatore Giacobbe, ho fatto parte del Comitato per le questioni degli italiani all'estero nella scorsa legislatura.

così come potremo garantire invece con l'impegno di tutta la Commissione affari esteri, emigrazione con l'indagine conoscitiva, a cui facevano cenno i colleghi e che ricordava il senatore Pellegrini, che andrà avanti per l'intera legislatura e che potrà

tutte le questioni che riguardano le comunità degli italiani nel mondo, le loro esigenze, i loro problemi e le loro rivendicazioni. Ricordo che c'è una grande novità in questa legislatura, che vede coinvolte le Commissioni affari esteri di Camera e Senato. Se ci fosse il presidente Casini potremmo chiedere a lui, che era presidente della Commissione affari esteri, emigrazione nella scorsa legislatura, quante volte abbia partecipato in cinque anni di legislatura ai lavori dell'Assemblea permanente del Consiglio generale degli italiani all'estero: zero. Dall'inizio di questa legislatura insieme naturalmente alla partecipazione dei senatori e dei deputati eletti all'estero, che non vedranno assolutamente intaccata la loro funzione, c'è una grande novità.

consumando italiano, dobbiamo garantire l'interesse di tutto il Senato della Repubblica e questo interesse lo possiamo suscitare se ad occuparsene sarà la Commissione affari esteri, emigrazione e non un Comitato autoreferenziale.

Me lo dicano i colleghi. Altri colleghi, giustamente, dicevano che negli anni non si è riusciti a far capire quanto sia importante il ruolo

M5S)*. Un percorso di cambiamento destinato a far crescere la visibilità di tutte le comunità del nostro Paese che vivono all'estero e soprattutto della consapevolezza di tutti i senatori, perché non vi sia un momento in cui un singolo organismo, composto soltanto da dieci senatori, possa occuparsi delle questioni rilevantissime che riguardano le nostre comunità. Voglio citarvi alcuni dati. Quanti in quest'Aula con il lavoro svolto dal Comitato in quattro legislature conoscono alcuni dati che riguardano i nostri concittadini all'estero.

le province del Sud Italia, ma sono, in ordine decrescente per numeri, Milano, Roma, Genova, Torino e Napoli. Le Regioni più coinvolte dai nuovi fenomeni migratori nell'arco del 2018, ancora una volta, non sono le solite Regioni del Sud o del Centro-Sud. La prima Regione di partenza è la Lombardia, con 22.000 persone andate via nel 2018,

conoscitiva che coinvolgerà tutti gli attori istituzionali, a partire dal Consiglio generale degli italiani all'estero, fino ad arrivare ai Comites, alle ambasciate, ai consolati

tema trattato in numerosissime sedute. Ricordo a tal proposito che la Commissione di cui mi onoro di far parte è stata l'unica Commissione e l'unico organo istituzionale nel Paese

di un decreto ministeriale che sarebbe dovuto intervenire sei mesi dopo l'approvazione della legge. Non è responsabilità di questo Governo; o meglio, a luglio non era responsabilità di questo Governo

vorrei che ci si concentrasse sugli effetti che dal 30 dicembre 2016 ad oggi sono scaturiti rispetto

e da soli, 14 o 15 persone su 315, hanno approvato una norma che si è insinuata nelle strade,

territorio, giovani, cultura della legalità, luoghi oscuri, impossibilità e incapacità da parte delle Forze dell'ordine di fermare un'*escalation* assurda, perché non esistono droghe leggere e droghe pesanti; esistono le droghe e questo è un altro concetto caro a tutti noi. Esistono le droghe e basta. Dovete sapere che nel 2017, quindi l'anno in cui il provvedimento è stato efficace, c'è stato l'11,5 per cento in più di sanzioni elevate dalle Forze dell'ordine per l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Dovete sapere che gli incidenti stradali con feriti e morti nell'anno 2017 sono stati 1690,

per cento di mortalità dovuta ad incidenti stradali, e tutti legati all'utilizzo di stupefacenti. Ora, la questione è, appunto, questa. Quello che noi oggi vogliamo capire nel dibattito parlamentare (e io spero che emerga anche, alla fine, nel voto finale) è se coloro i quali non hanno partecipato a questo disastro legislativo e che oggi potrebbero avere i numeri per poter ribaltare il risultato hanno la voglia di farlo. C'è la voglia di farlo? Io spero anche in coloro i quali all'epoca l'hanno sostenuta perché, quando il Governo uscente, quindi precedente a questo, prima di andare via, attraverso la figura del segretario generale del Ministero della salute, chiese al Consiglio superiore di sanità un punto di vista, un parere, sulla commercializzazione e l'utilizzo della cosiddetta *cannabis*, anche in percentuale ridotta (la cosiddetta *cannabis* *light*), il Consiglio superiore di sanità dette delle risposte lapidarie.

tale consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e quindi gli effetti psicotropi che questi possono produrre, sia a breve che a lungo termine sono pericolosi;

ritenendo, relativamente alla questione dell'utilizzo delle cosiddette infiorescenze di *cannabis* che: «in forza del parere sopra espresso circa la loro pericolosità, qualunque ne sia il contenuto percentuale, pone certamente motivo di preoccupazione e raccomanda che siano attivate, nell'interesse della salute individuale pubblica, in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti». Ebbene, invece, cosa succede? Che ad ogni angolo di strada abbiamo quelli che, probabilmente, nel Nord Europa si chiamano *coffee shop*. Abbiamo luoghi in cui si vende la *cannabis light* in ogni bevanda, nei prodotti, nelle caramelle, nei dolcetti.

Affoga questi dispiaceri in una praticità di recupero di sostanze stupefacenti. Concludo, Presidente, chiedendo un impegno del Governo - e spero di tutti i colleghi che si ritengono contro la legalizzazione della droga - ad emanare urgentemente, a seguito di un parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, un provvedimento per la sospensione immediata della commercializzazione di tutti i prodotti e della cosiddetta *cannabis* *light*; ad attivarsi con urgenza prevedendo una regolamentazione più stringente delle modalità di coltivazione e commercializzazione della canapa; a valutare l'opportunità di destinare in altro modo le risorse economiche di cui al comma 1 - perché gli diamo anche 700.000 l'anno a questi per andare a fare drogare i nostri figlioli e ad emanare urgentemente un decreto ministeriale, come prescritto dall'articolo 5 della citata legge, per definire i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti; a verificare se le condotte della addirittura nota come Cannabis business school siano conformi alle prescrizioni di legge. Insomma, in una parola: chi è a favore delle droghe voti contro; chi è contrario voti a favore della nostra mozione.

Signor Presidente, anzitutto una battuta: credo che il senatore Mallegni abbia sbagliato legge; probabilmente si è confuso e ne ha letta un'altra. 242 del 12 febbraio 2016, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, prevede tra le proprie finalità il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. La legge sostiene e promuove la coltivazione, la trasformazione e lo sviluppo delle filiere finalizzate alla produzione di prodotti tessili, di semilavorati da impiegare nella bioedilizia, nella componentistica, di prodotti alimentari (principalmente semi, oli e farina). Se l'utilizzo della canapa quale prodotto tessile appare piuttosto problematico per gli alti costi, altri settori risultano particolarmente interessanti per le prospettive di realizzazione di margini economici rilevanti, che permetterebbero all'agricoltore di ottenere prezzi superiori per la materia prima rispetto a quelli attualmente riconosciuti ad altre produzioni. La legge non prevede, tuttavia, l'istituzione del tavolo di filiera che, come avviene per altre colture, ha il compito di definire le attività da intraprendere per il sostegno del settore, a partire da un'analisi del comparto che ne metta in luce le potenzialità e i punti di debolezza, individuando le linee di ricerca che risulta più urgente perseguire, favorendo lo scambio di informazioni di natura tecnica e scientifica, indirizzando al contempo l'utilizzo delle risorse a disposizione. Il sostegno al settore della canapicoltura e alla strutturazione delle filiere si sostanzia nella norma finanziaria prevista dall'articolo 6 della legge, agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa e una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'agricoltura, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Considerato che attualmente, in Italia, i negozi *grow shop* dedicati alla vendita della canapa con bassi livelli di THC e prodotti derivati sono più di 400 ricordando che l'articolo 18*-quater* del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile, la rimborsabilità è a carico del Servizio sanitario nazionale ed è subordinata alle indicazioni delle singole Regioni;

al fine di consentire alle persone malate di questo Paese il diritto all'uso terapeutico della cannabis; considerato infine che è compito di un Paese civile dare risposta ai problemi con la certezza della scienza e senza i falsi timori derivanti da pregiudizi senza alcun fondamento scientifico, impegna

ad assumere le iniziative necessarie al fine di provvedere alla riorganizzazione organica della materia relativa alla filiera agroindustriale della canapa per garantire a tutti gli operatori del settore una normativa certa cui attenersi, nonché ad adottare le iniziative necessarie a confutare falsi timori in materia, derivanti da pregiudizi senza alcun 2) a definire, con decreto del Ministero della salute, i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti così come previsto dall'articolo 5 della legge n. 242 del 2016, ponendo così fine ai margini di incertezza per un compiuto inquadramento della tematica; 3) ad adottare ogni iniziativa utile alla costituzione ufficiale del tavolo di filiera al fine di favorire il reale sviluppo di intese sia per quanto riguarda le produzioni alimentari, sia quelle tessili, sia quelle impiegate nel settore della bioingegneria; bioingegneria; 4) ad adottare ogni iniziativa finalizzata all'assegnazione delle risorse individuate dalla legge n. 242 del 2016 alle finalità dalla stessa indicate.

il Consiglio superiore di sanità, che poi è stato smobilitato, aveva rilevato la pericolosità anche della cosiddetta *cannabis light*. Colleghi, qui si parte - a volte - da aspetti agricoli e produttivi,

delle conseguenze negative e oggi il proliferare di negozi e negozietti è quasi un'azione di propaganda e promozione della legalizzazione. Vi siete chiesti come mai, negli ultimi anni,

Non sottovaluto altre forme di dipendenza: l'alcol, ad esempio, ma oggi anche la ludopatia è un fenomeno che ha avuto dimensioni sociali preoccupanti. Ma rimanendo sul tema delle dipendenze da sostanze stupefacenti, vorrei invitare il Governo a non limitarsi a un'intervista periodica o alla proposta di legge. Giustissimo: lo spacciatore va punito. Anch'io ho letto con raccapriccio le notizie che sono giunte da Porto Recanati, giorni fa, di una persona straniera - ma lasciamo perdere se straniera o italiana, poteva succedere a persone di qualsiasi nazionalità - che, andando contromano con l'automobile, ha ucciso due giovani genitori che lasciano due bambini. E poi si scopre che questa persona era stata arrestata, poi evidentemente liberata,

che hanno i grandi spacciatori, che poi diventano, sulle strade, *killer* di famiglie: c'è una connessione. Ho visto che giorni fa, ad esempio, il congresso di Magistratura democratica

perché alcune norme sono state cassate. Ad esempio, c'era la dose media giornaliera, che era quella al di sopra della quale una persona si poteva considerare spacciatore e non consumatore, laddove il consumatore va recuperato alla vita civile, non è che deve essere sbattuto in carcere,

Il Dipartimento per le dipendenze, che aveva avuto stagioni importanti con Governi di centrodestra, è inerte e inattivo. Quindi, come vedete, noi riproponiamo una politica di prevenzione, di informazione corretta sulle sostanze e sui loro pericoli, anche della *cannabis light*, anche dei negozietti. Invece c'è una grande sottovalutazione. Giorni fa anche il ministro Salvini, illustrando la proposta di inasprimento delle sanzioni, ha detto: «però non voglio andarne a parlare nelle scuole». Invece, è nelle scuole che dobbiamo parlare dei pericoli delle droghe, in maniera educativa

prodotte e gestite in un circuito molto preciso. Anche l'Istituto farmaceutico militare, che sta a Firenze, si occupa della produzione di *cannabis* ai fini terapeutici, in una situazione di controllo (ammesso che poi siano utili, ma di farmaci ce ne sono tanti). Noi temiamo coloro che, non sapendo nulla di medicina, parlano degli effetti positivi terapeutici della *cannabis* perché puntano e legalizzarla e a farla consumare in maniera irresponsabile soprattutto dai nostri minorenni. *(Applausi dal per ricordare che anche le battaglie sulla legalizzazione non servono a nulla. Si dice che così si sconfigge il crimine: colleghi, per la criminalità, i proventi delle cosiddette droghe leggere rappresentano una quota minimale dei loro profitti. I soldi li fanno con l'eroina, con la cocaina, con le droghe chimiche. Anche se si legalizzassero le cosiddette droghe leggere termine che io non accetto - andremmo a scalfire una piccola percentuale e siccome di quella piccola percentuale tre quarti dei consumatori - ahimè - sono minorenni, ai quali non si potrebbe somministrare la droga legale (in teoria, nemmeno le sigarette potrebbero comprare dal tabaccaio senza dimostrare di essere maggiorenni), noi non scalfiremmo in alcun modo i proventi della criminalità, come ha spiegato Gratteri, un importante procuratore della Repubblica, che ha combattuto e combatte il narcotraffico. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. La mozione ci consente di ridiscutere di tutte queste cose. condivido le parti dispositive della mozione, che parlano del decreto ministeriale per definire i livelli massimi di residui di THC (tetraidrocannabinolo), per evitare una cultura minimalista del negozio della porta accanto. Se quella *light* la vendono sotto casa, non farà poi tanto male:

avere una assuefazione. Dico anche al Governo di occuparsi della Conferenza nazionale, del dipartimento messo in sonno e anche di un'informazione corretta sui pericoli delle droghe e sostenere le comunità terapeutiche, perché noi che siamo contro la legalizzazione delle droghe siamo, non a caso, i più grandi sostenitori di chi recupera i tossicodipendenti, ai quali non va data droga legale (*cannabis* *light* o non so che cosa) ma va data un'alternativa di vita, dal Gruppo FI-BP)*. Se poi oggi quelle comunità, laiche o religiose, di varia natura e tipo, sono state contrastate, è inutile lamentarsi che non c'è chi tende una mano, perché nei SERT, con tutto il rispetto per gli operatori pubblici, danno un po' di metadone, non danno un aiuto. Questa mozione, che introduce alcune considerazioni giuste sul THC, sull'uso e sull'abuso della canapa, sul tema della *cannabis light*, su negozi e negozietti, credo che sia un'occasione per invitare il Governo (le mozioni sono anche atti d'indirizzo) a riprendere una forte iniziativa. Vanno bene gli annunci di una proposta di legge e le interviste periodiche,

le sue proposte concrete, ma soprattutto come momento di riflessione del Parlamento per combattere le droghe, tutte le droghe, con la solidarietà, con la vita, con l'educazione. Lo spaccio va represso, ma la dipendenza va contrastata con valori e un'educazione sana.

Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, già oggi la normativa vigente prevede regole molto stringenti per quello che riguarda l'utilizzo della canapa e la sua commercializzazione. Il commercio delle infiorescenze (e in genere dei prodotti derivanti dalla canapa) deve ritenersi consentito se il contenuto di THC non supera il limite dello 0,6 fissato dall'articolo 4 della legge n. 242 del 2016 in riferimento alla coltivazione della canapa. Ad oggi, superato tale limite,

In particolare la III sezione penale della Cassazione lo scorso 6 dicembre 2018 ha confermato che la legge n. 242 del 2016 consente la commercializzazione dei prodotti della coltivazione della canapa ma a tre condizioni. La prima è che deve trattarsi di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC. è che la percentuale di THC presente nella canapa non deve essere superiore allo 0,2 per cento. La terza è che la coltivazione deve essere finalizzata alla realizzazione di una serie di prodotti espressamente e tassativamente indicati nella stessa legge. Va detto che, allo stato attuale, la *cannabis light* (intesa come infiorescenze) e i prodotti da essa derivati non dispongono di una norma specifica che obblighi le infiorescenze e i prodotti derivati a rispettare criteri di sicurezza e qualità se consumati ad uso umano. Pur rispettando il limite dello 0,2 per cento infatti, questi prodotti non godono di una normativa *ad hoc* per la realizzazione di prodotti destinati al consumo umano, né rientrano nella categoria degli integratori o degli alimenti, la cui liceità o meno non è chiara ed è lasciata ad interpretazioni personali e restrittive. Ecco perché questi prodotti ricorrono all'*escamotage* dell'uso tecnico o collezionistico per giustificarne la vendita, indipendentemente dal contenuto in metalli pesanti, pesticidi, aflatossine, muffe e batteri, anche se di fatto il consumatore a casa è libero di fumarla, vaporizzarla, utilizzarla come ingrediente alimentare o per preparare estratti. Rischi concreti per la salute ci sono. E gli estratti da infiorescenza, è indubbio, consentono di ottenere prodotti finali che, da uno 0,6 per cento di partenza nel fiore, possono arrivare a contenere il 2, il 3, il 4 e fino al 5 per cento di THC nell'estratto finito, a seconda della quantità di infiorescenza e del metodo di estrazione utilizzato. Qui però evidenzio e voglio porre l'attenzione sul fatto che non viene centrato il cuore del problema, cioè la possibilità dell'uso terapeutico della *cannabis*. Purtroppo, nel sapere comune, si tende ad unificare delle realtà che niente hanno a che vedere l'una con l'altra. La *cannabis* terapeutica o medica - settore che andrebbe incentivato - nulla ha a che vedere con la canapa della legge n. per diversità di genetica, di tecniche di coltivazione, di contenuto in THC e CBD e per gli stessi controlli obbligatori di un farmaco industriale. In Italia, la *cannabis* medica è stata autorizzata come sostanza da utilizzare nelle preparazioni galeniche eseguite in farmacia dal 2013; in seguito, nel 2015, ne è stata normata la produzione, la vendita e la distribuzione.

Sebbene il mercato permetta di averne a disposizione molta di più, si assiste a una cronica carenza di *cannabis* terapeutica. Le quantità disponibili annualmente sono inferiori anche alle sole richieste delle prescrizioni mediche. Nel tentativo di arginare il problema, nel novembre 2017 il Ministero della salute, insieme a quello della difesa, hanno avviato un bando per l'importazione di ulteriore *cannabis* medica, che ad oggi si è comunque dimostrato insufficiente. Vi è un pregiudizio culturale, dovuto in massima parte a disinformazione, che si concretizza con attività che danneggiano ulteriormente chi, in maniera professionale, si adopera per fornire ai pazienti queste tipologie di medicinali: le principali farmacie italiane che preparano *cannabis* terapeutica ai pazienti sono da anni soggette a controlli eccezionali da parte di AUSL, NAS e AIFA. La facoltà del Ministero della salute di effettuare rigorosi controlli non può essere messa in discussione, anche se in passato tutto ciò si è tradotto in rallentamenti nelle forniture e in pendolarismo dei pazienti alla ricerca della farmacia con il prodotto disponibile, ma anche nella rinuncia di nuove farmacie alla preparazione delle terapie a base di *cannabis*. Anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha rilasciato uno *statement* in cui raccomanda la riclassificazione della *cannabis* come farmaco, indicando di escludere dalle droghe i prodotti che contengono THC in misura inferiore allo 0,2 per cento, ritenendoli non stupefacenti. Concludo con l'auspicio che anche l'Italia, proprio per rispondere alle esigenze di quei pazienti con patologie molto dolorose, sblocchi definitivamente il problema dell'approvvigionamento della *cannabis* terapeutica, lasciandola esclusivamente alla prescrizione del medico e alla preparazione del farmacista. Grazie

le mozioni poste oggi in discussione hanno sollecitato un dibattito su un tema particolarmente complesso. È doveroso premettere esse non consentono l'assunzione di impegni definitivi da parte del Governo, in assenza dei necessari approfondimenti sia di natura giuridica che scientifica, i quali non a caso, per quanto siano stati avviati già sul finire della scorsa legislatura, non sono tuttora pervenuti a una univoca conclusione. Bisogna dire effettivamente che esiste una certa difformità giuridica, facilmente verificabile dalle sentenze attualmente disponibili, così come esiste anche una carenza di dati scientifici. Ho sentito dagli illustri senatori diversi spunti positivi in proposito, anche altamente condivisibili. Mi si consenta, però, di fare una piccola precisazione, soprattutto rispetto a quanto esposto dal senatore Gasparri. Al di là di alcune affermazioni, che possono essere in parte condivisibili, mi è sembrato di percepire una sorta di messaggio un po' distorto che riguarda, per esempio, il giudizio del precedente Consiglio superiore di sanità che, a detta dello stesso, forse sarebbe stato dismesso appunto per il parere sulla canapa. Questa è una cosa che mi lascia un po' perplesso, perché equivale a dire che il gruppo di scienziati arruolati oggi nel Consiglio superiore di sanità sono verosimilmente tutti proni all'uso della *cannabis.* Tranquillizzo quindi il senatore Gasparri che personalmente di far fare l'analisi del capello a tutti i componenti del Consiglio superiore di sanità, qualora fosse necessario. In ogni caso, in ragione dell'alta considerazione che il Governo assegna agli impegni assunti in questa sede, dico subito che la complessità della disciplina introdotta con la legge n. 242 del 2016 - sulla cui applicazione faccio notare che non è stata raggiunta nemmeno unanime condivisione a livello giurisprudenziale e la presenza, inoltre, di numerosi e rilevanti profili che coinvolgono una pluralità di amministrazioni, sono tutte circostanze che non consentono di esprimere un avviso definitivo, che rischierebbe solo di semplificare e banalizzare la molteplicità di aspetti, che, ripeto, sono sia di natura giuridica che scientifica.

possono essere utilizzati come fumo, per cui rientrerebbero nella legislazione riguardante il tabacco. Non ultima, la problematica della *cannabis* ad uso terapeutico, che non è stata menzionata in queste mozioni, ma che sicuramente è un altro aspetto importante da trattare, per cui il tema è estremamente complesso. Dalle attività condotte dal Ministero della salute emerge dunque, innanzitutto, che i possibili rischi per la salute risiedono in un abuso nell'elusione della disciplina vigente e, pertanto, in un profilo patologico delle condotte concretamente messe in pratica, per quanto esse invochino un'asserita aderenza alla legislazione vigente. peraltro, che nell'esercizio delle proprie competenze il Ministero dell'interno ha provveduto in più occasioni - da ultimo con circolare del 15 gennaio 2019 - a dare indicazioni operative alle Forze dell'ordine e alle Forze di polizia che, pur tenendo conto del complesso quadro della materia, hanno fornito un indirizzo nelle attività di controllo e contrasto alle condotte non conformi alla legge. Tutto ciò premesso, nel ribadire che la valutazione del Governo non può che essere negativa sul complesso delle mozioni presentate, a riprova della serietà dell'attività che si intende svolgere nella materia oggetto di discussione, si ritiene di poter accogliere taluni impegni, come di seguito specificati.

Sull'impegno 2) il parere è favorevole, a condizione che venga così riformulato: «a valutare l'opportunità, in esito ai necessari approfondimenti, sia di natura giuridica che scientifica, peraltro già in atto, di prevedere una nuova regolamentazione delle modalità di coltivazione e commercializzazione della canapa». Sull'impegno 3) il parere è favorevole a condizione che venga così riformulato: «a valutare l'opportunità di destinare le risorse economiche di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 242 del 2016 anche per altre finalità, tra cui la ricerca».

«a valutare l'opportunità, in esito ai necessari approfondimenti sia di natura giuridica che scientifica, peraltro già in atto, di prevedere una nuova regolamentazione delle modalità di coltivazione e commercializzazione della canapa».

«a valutare l'opportunità di destinare le risorse economiche, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, anche per altre finalità, tra cui la ricerca».

svuotino di significato il nostro punto di vista. Solo per cercare di argomentare e essere conseguentemente cortesi rispetto all'impegno che il Governo ha messo nella riformulazione, al punto 2), dove si chiede di «valutare l'opportunità, in esito ai necessari approfondimenti sia di natura giuridica che scientifica, peraltro già in atto, di prevedere una nuova regolamentazione delle modalità di coltivazione e

normativa carente perché mancante di un provvedimento significativo del Ministero, e potrebbe dare una mano a tutto il territorio. Senatore Mallegni, l'opportunità c'è, a condizione che l'Assemblea concordi sul fatto di votare per parti separate.

Sono fortemente dispiaciuto di non poter esprimere singolarmente il punto di vista, perché avrebbe potuto essere costruttivo; di conseguenza, non posso far altro che prendere atto di un diniego che ovviamente corrisponde ad un ulteriore diniego da parte nostra.

avremmo preferito che ci fosse stata una discussione complessiva sul problema delle droghe in Italia. Avevamo chiesto, in Conferenza dei Capigruppo, che fosse calendarizzata anche una mozione di Fratelli d'Italia che era stata presentata nel mese di giugno del 2018, proprio per fare in modo che la discussione non vertesse esclusivamente su aspetti parziali, perché siamo al cospetto di una vera e propria emergenza nazionale. Lo dicono i dati che vengono diffusi in maniera ufficiale: un terzo della popolazione compresa nella fascia di età tra i quindici e i ha fatto uso di droghe almeno una volta nella vita. Una percentuale che arriva addirittura al 43 per cento se si considera la fascia di età tra i quindici e i

Non meno preoccupanti sono i dati circa il fenomeno della tossicodipendenza in termini di persone denunciate; un aumento nel decennio 2007-2017 di oltre il 6 per cento, con un aumento delle operazioni antidroga delle Forze dell'ordine che ha superato il 21 I dati relativi ai sequestri vedono un aumento dei quantitativi di cocaina del 55

per quanto riguarda la *marijuana*, addirittura del 963,6 Sono dati che la dicono tutta sulla preoccupazione che ognuno di noi deve vivere voglio ricordare, come ha già fatto il senatore Gasparri, che la Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti si è tenuta l'ultima volta a Trieste nell'ormai lontano 2009. Abbiamo inoltre costituito presso la Presidenza del Consiglio un Osservatorio permanente dal dicembre del 2017, ma non abbiamo traccia alcuna della sua attività. Questo per dire che certamente gli aspetti oggi in discussione sono importanti e voglio dichiarare a nome del Gruppo Fratelli d'Italia

abbiamo il dovere, al di là dei modelli ideologici, di mettere al primo posto la salute dei nostri cittadini e, in particolare, dei nostri giovani. Non sottaciamo neanche il fatto che noi crediamo che un'ulteriore spinta al modello di deresponsabilizzazione sociale, della droga a portata di mano seppur con un THC depotenziato rappresenti, in particolare per i nostri giovani, un'altra occasione deleteria per indirizzare le proprie vite. La droga ha effetti distruttivi sulle capacità mentali dell'uomo ed effetti

ma pensiamo che ci sia bisogno di un'azione di carattere culturale, che vada ad incidere sulla vita sociale, proponendo un modello che rifiuti la droga. C'è bisogno di azioni, c'è bisogno del racconto delle esperienze di chi ha vissuto l'errore di coloro che lavorano in questo settore e sono impegnati nel recupero, c'è bisogno di un'azione all'interno delle nostre scuole, per dire ai nostri ragazzi che la trasgressione non è questo, questo è soltanto un danno alla salute. Oggi essere anticonformisti e trasgressivi significa essere impegnati per dare uno sfogo positivo al proprio cervello, per dare uno sfogo in termini di impegno culturale, di impegno sociale nel volontariato e magari nella più alta forma di passione civile, che è la politica, per migliorare la nostra Patria e quindi Ci aspettiamo dal Governo un impegno forte in questo senso, ma anche concreto, perché la repressione è certamente l'antibiotico necessario alla febbre, ma c'è bisogno di un vaccino, ovvero di promuovere e rinforzare il sistema di monitoraggio, di promuovere campagne informative efficaci soprattutto tra i più giovani e di rinforzare con urgenza il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con la destinazione di almeno 50 milioni milioni di euro, e di ampliare i compiti del Dipartimento per le politiche antidroga, proprio per realizzare un'azione di contrasto che sia sinergica.

dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, che provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali, a base di *cannabis*, per la successiva distribuzione alle farmacie, che la dispensano dietro ricetta medica non ripetibile, la rimborsabilità è a carico del Servizio sanitario nazionale ed è subordinata alle indicazioni delle singole Regioni. Tra le altre cose, lo stabilimento di Firenze ha anche la facoltà di svolgere studi clinici in materia. sede si è invece parlato della *cannabis* ricreativa, che è un'altra cosa e che ha un principio attivo (il famoso THC) superiore a quello di cui stiamo parlando adesso e quindi di quello citato nella legge n. 242 del 2016, che riguarda la produzione agroalimentare.

ha sperato e spera ancora in una giusta rivalutazione di una coltura che nel passato è stata una delle voci principali dell'economia di vaste aree di alcune Regioni del nostro Paese. La normativa interessa una molteplicità di settori relativi alla coltivazione, alla trasformazione e alla incentivazione dell'impiego e del consumo finale dei semilavorati provenienti dalle filiere locali, allo sviluppo di filiere territoriali che valorizzano la ricerca, l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica dei semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori

risposta a un settore che è andato in crisi a causa dell'inaccettabile e strumentale accostamento alla più famosa canapa indiana, dell'intensità del lavoro e anche della competizione, proveniente in special modo dagli Stati Uniti, di fibre sintetiche meno costose e più moderne. Non tutti forse sanno che con la canapa si può fare anche la carta, si possono fare tessuti, corde, oli, medicine; si può utilizzare come combustibile e probabilmente lo sviluppo di questo comparto rappresenta un problema per per tutti quei settori che si sono arricchiti e che continuano a farlo inquinando con plastica e petrolio. Nonostante il lungo periodo di blocco della produzione - parlo sempre di quella agroalimentare ovviamente - causato dalle politiche proibizionistiche, oggi l'aumento continuo del prezzo del petrolio e la crescente attenzione per la tutela dell'ambiente hanno comportato una ripresa della coltivazione e produzione della canapa industriale in molti Paesi europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Polonia e Romania (quindi non siamo da soli). Credo che, come è stato fatto in quest'Aula, occorra avere un approccio diverso rispetto a questo tema ed uscire dagli schemi mentali troppo ideologici. Abbiamo parlato di droghe e dei nostri ragazzi; abbiamo parlato di

che ne metta in luce le potenzialità e i punti di debolezza. Forse, in questo modo sarebbe stata favorita una riflessione differente e lo si poteva fare anche oggi in Assemblea. Della *cannabis* terapeutica vi ho già parlato. È molto importante, noi lo sappiamo e stiamo sostenendo anche delle leggi a favore di chi ha problemi

positivi. Come si può evincere, non c'è quindi bisogno di creare allarmismi; non si sta parlando di liberalizzazione, ma di regolamentare e applicare la normativa esistente. Ricordo che l'Organizzazione mondiale della sanità ha richiesto la rimozione della *cannabis* dalle liste delle sostanze più pericolose, riconoscendo quindi legittimo l'uso terapeutico di *cannabis* e cannabinoidi, in contrasto con la posizione del 1954 che incitava a compiere sforzi verso l'abolizione della *cannabis*

A questo punto, credo che davvero sia compito del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, perché stiamo parlando di queste due leggi importanti, effettuare ulteriori studi e approfondimenti per confutare falsi timori in materia, derivanti da pregiudizi senza alcun fondamento

ponendo così fine ai margini di incertezza per un compiuto inquadramento della tematica. Quindi, è questo che vogliamo: regolamentare dove è giusto che sia. Le leggi ci sono, le dobbiamo rendere attive e chiediamo un impegno al Governo per questo.

onorevoli senatori, membri del Governo, noi pensiamo invece che non ci sia confusione su questa tematica e che sia tutto molto chiaro. Siamo di fronte a due mozioni che vogliono, sì, regolamentare il settore,

confutare falsi timori in materia derivanti da pregiudizi senza alcun fondamento scientifico. Quindi, è tutto molto chiaro per quanto ci riguarda. Così come, pur apprezzando

sempre che ci siano poi delle proposte che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra. Riteniamo che le Commissioni debbano poter adottare, verificare, studiare e fare tutte le audizioni possibili, ma che non si possa possa prendere una decisione in questa sede. Anche perché, se è compito del Parlamento, poi impegniamo il Governo? Ma che sia il Parlamento, eventualmente, se ha i numeri e la forza, ad andare in una direzione piuttosto che in un'altra oppure a lasciare tutto com'è. Motivo questo visto che non è questa la sede, voteremo contro sia alla mozione n. 31, presentata da Forza Italia, che alla mozione n. 89, presentata dal Partito Governo, mi associo alla premessa che ha fatto la collega Boldrini

un minimo il "filo storico" di queste leggi. Mi riferisco alle ultime legislature. Intanto, l'attenzione che il Parlamento ha sempre avuto nei confronti della *cannabis* terapeutica

proprio perché il paziente non dovesse andare con la fotocopia della ricetta a farsene fare un'altra per poter avere i farmaci di cui aveva bisogno per affrontare la sua situazione, con tutto il dolore e la sofferenza che comporta.

le patologie di tipo contratturante e alcune forme di epilessia. Queste sono le indicazioni terapeutiche di elezione della *cannabis*. Ma non è di questo che stiamo parlando,

Voglio, però, ricordare che nell'ultima legislatura la norma sulla *cannabis* terapeutica è stata stralciata da una legge che in realtà prevedeva la liberalizzazione dell'uso della *cannabis*. Soltanto l'idea di ricondurne l'uso all'esclusivo fine terapeutico permise l'approvazione della legge in Aula, altrimenti nel dibattito che ne sarebbe nato l'opposizione sarebbe stata molto forte e molto intensa. Voglio dire che noi qui ne stiamo parlando oggi non perché ci preoccupiamo degli usi, per esempio, come combustibile o per i tessuti: siamo tutti d'accordo che quella filiera agroalimentare possa avere tutta la sua ragione di esistere. Qui stiamo parlando della *cannabis* perché assumiamo una responsabilità precisa, forte e concreta nei confronti di coloro che, facendo uso di *cannabis*,

è vero che non tutti coloro che, come si dice in gergo, si fanno uno spinello poi diventano dipendenti; siamo tutti d'accordo, ma è vero anche il contrario: tutti coloro che ne diventano dipendenti hanno cominciato con lo spinello. *(Applausi

sanità, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche e una serie di esperti nazionali del Punto focale. Signori, se me lo permettete, poiché è una cosa semplicissima,

che ho semplicemente copiato da quella relazione. L'autorevolezza di quanto vi dico non deriva da me e neanche, se volete, da un'esperienza maturata in quarant'anni di onesto lavoro come neuropsichiatra infantile. No, deriva dai numeri che diversi Ministeri ci hanno trasmesso nella loro relazione al Parlamento. Sono a disposizione di tutti e sono numeri, cifre, dati che non possono non preoccuparci.; prima di tutto perché il consumo di *cannabis* è cresciuto (un ragazzo su tre),

e ci dice proprio questo. Ci dice che molto spesso l'uso della droga - anche della *cannabis* - non è isolato. Spesso chi fa uso di *cannabis*,

Signori, sappiamo perfettamente cosa succede in tante discoteche, non possiamo nasconderci. Sappiamo - si tratta di dati in circolazione in questi giorni - che una forma di *cannabis* sintetica a bassissimo costo sta

Sappiamo che c'è una furbizia diabolica che mette queste persone nella condizione di avvicinarsi e approssimarsi sempre di più a questo consumo.

cosa. Sappiamo che è in aumento il numero delle persone che cercano di essere accolte nelle comunità e sappiamo quanto sia difficile, se queste comunità non dispongono di risorse economiche e personale qualificato, che le persone realmente ne escano fuori.

allora riduciamo, togliamo, aboliamo, svuotiamo le nostre carceri, mandando questi ragazzi fuori». Sono d'accordo che il carcere non cura e non riabilita.

fu assegnato a una donna per una bellissima storia, dal titolo «Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio», in cui si racconta tutto un itinerario

emotivo" - così è definito - che avvicina i ragazzi problematici. Ci sono anche dei *test* che vengono fatti per individuare quali sono i ragazzi a più alto indice di rischio. Signori, noi stiamo parlando di questo: stiamo parlando di questo: della proliferazione che c'è stata - io dico a Roma, ma mi si dice in Italia - di negozi in cui è possibile comprare droga teoricamente a bassissima concentrazione. Di fatto, questi negozi si sono moltiplicati e non ci sono adeguati controlli. È sorprendente. Qual è l'elemento più pericoloso di questi negozi?

Non toglieteci la responsabilità di fare una forte azione di prevenzione; non trattateci da persone che non si rendono conto. Non siamo proibizionisti di non so che cosa: siamo educatori responsabili e consapevoli nei confronti delle future generazioni.

mi pare che si sia fatta un po' di confusione nell'esame di queste due mozioni, perché la canapa o *cannabis* è una pianta dalle molteplici funzioni e funzionalità, ed è una pianta della quale non si butta via niente. La legge n. 242 del 2016 ha cercato di normare, come primo passo,

È una pianta che certamente va rivalutata al di là di ogni fuorviante pregiudizio. Era utilizzata già per costruire cordami, tele per navi, carta e per estrarre essenze per fini medici. Diffusissima nel Nord America, ma anche in Italia (fino al secolo scorso), Paese che fu grande esportatore di fibre verso le varie marinerie d'Europa. Poi, circa un secolo fa, in epoca di proibizionismo, fu messa al bando col pretesto delle intrinseche proprietà psicotrope ed iniziò così il suo declino. però l'Organizzazione mondiale della sanità, dopo accurate valutazioni, ha raccomandato di togliere l'intera pianta di *cannabis* dalla tabella IV delle sostanze pericolose della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, ovvero da quella tabella che contiene le sostanze dannose e di valore medico e terapeutico estremamente ridotto.

Ma è opportuno distinguere la canapa o *cannabis light,* contemplata dalla legge n. 242 del 2016, dalla *cannabis* che definiamo medica, utilizzata e coltivata per fini farmaceutici. La pianta della canapa è utile per produrre fibre naturali, farina, oli, birra, cosmetici e farmaci naturali. È altresì in grado di rilasciare un considerevole quantitativo di materiale organico nel suolo, aumentandone la fertilità, ed è anche di contrasto alla desertificazione e alla perdita di biodiversità. Può essere assai utile nella rotazione colturale; si presta molto facilmente al metodo biologico ed è da considerarsi una grande risorsa in termini di bioeconomia circolare. L'interesse più recente per le piante da fibra in genere, e per la canapa in particolare, è dovuto fondamentalmente all'opportunità di riuscire a realizzare biomateriali per diverse tipologie di manufatti, sostituendo così le fibre sintetiche. Sotto il profilo commerciale è importante evidenziare che il fenomeno della vendita di prodotti derivanti dalla canapa industriale si è velocemente diffuso in Italia, unitamente al crescente interesse per i cannabinoidi non psicoattivi quali, ad esempio, il cannabidiolo (CDB) utilizzato per prodotti cosmetici. Sul tema, come già qualcuno ha avuto modo di esporre, si è espressa una recente sentenza della Corte di cassazione (sezione VI penale, n. 4920 del 2019) che ha stabilito che dalla liceità della coltivazione della *cannabis*, così come previsto dalla legge n. 242 del 2016, derivi anche la liceità della diffusione dei suoi prodotti contenenti il principio attivo THC in misura inferiore allo 0,6 cento. Nel senso che i prodotti con THC inferiore allo 0,6 per cento non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici), sostanze stupefacenti. Sempre questa pronuncia ha stabilito la valenza del principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell'ambito del generale potere delle persone di agire per il soddisfacimento dei propri interessi. Il MoVimento 5 Stelle conosce bene la tematica e, già durante la scorsa legislatura, ha promosso il rilancio della filiera della canapa con azioni concrete e con l'avanzamento di una proposta poi diventata legge. Mi riferisco alla già citata legge n. 242 del 2016, che nasce per mettere le basi per un importante comparto dell'economia agricola. La coltivazione di tale pianta, che avrebbe dovuto determinare una delle possibilità di crescita del settore, purtroppo, è stata arrestata a causa di aspetti determinanti non regolati dalla stessa legge. Di recente, la comunità scientifica ha posto sempre più attenzione al possibile impiego dei diversi principi attivi derivanti dalla *cannabis* medica, fra i più importanti: il cannabidiolo (CBD), sostanza non riconosciuta come psicotropa, ed il tetraidrocannabinolo (THC), sostanza psicotropa, da destinare a molteplici finalità terapeutiche. Nella letteratura scientifica si trovano innumerevoli ricerche volte a testimoniare gli enormi benefici riscontrati dall'impiego dei principi attivi; questi studi ed il crescente interesse della ricerca lasciano intendere come tali derivati possano in un prossimo futuro assumere una grande rilevanza e valenza per le scienze farmacologiche. Attualmente in Italia è consentito, a persone che possiedono una prescrizione medica, acquistare tali sostanze presso le farmacie che dispensano la *cannabis* ad elevato tenore di THC. Molti farmacisti eseguono tali preparazioni galeniche nel rispetto della normativa vigente, seguendo le indicazioni riportate nella prescrizione medica che riporta il valore di THC da conferire alla preparazione, partendo dalla materia grezza (infiorescenze essiccate di *cannabis* medica) reperibile sul mercato farmaceutico e acquistata dalle farmacie che ne hanno fatto richiesta. Secondo norma, tale preparazione deve essere fatta con procedura estemporanea e *ad personam* e non può, quindi, essere preparata in lotti. Procedura pertanto già assai farraginosa. Solo una parte del fabbisogno interno viene soddisfatta dall'Istituto farmaceutico militare di Firenze, che non riesce a soddisfare le richieste di una domanda interna in continua crescita. Il resto della *cannabis* ad uso medico proviene dall'estero secondo canali ufficiali ed i prezzi per i pazienti raggiungono anche valori proibitivi. A questo punto, si rende evidente la necessità di reperire possibilmente in Italia la materia prima e di snellire le procedure di preparazione galenica ad uso terapeutico. Inutile celare la possibilità che oggi, attraverso Internet e in un mondo sempre più globalizzato, chiunque possa aggirare regolamenti e norme e farlo molto facilmente. Sarebbe auspicabile promuovere la ricerca per riuscire a estrarre e separare dalla canapa industriale tali principi attivi, ciò previo un rigoroso controllo, così da ottenere un aumento della produzione che porterebbe a un auspicato abbassamento dei prezzi. Tale procedura potrebbe mettere il nostro Paese in linea con altri Paesi europei e con gli Stati Uniti e il Canada, che stanno investendo molto in ricerca su questi nuovi farmaci e sull'estrazione dei cannabinoidi da materiale grezzo. da materiale grezzo. La possibilità di estrarre tali principi attivi da poter impiegare in campo farmaceutico potrebbe rilanciare l'interesse verso la coltivazione della canapa industriale a pieno campo, nel rispetto della attuale normativa di riferimento e favorire l'apertura di centri di lavorazione sul nostro territorio, con conseguente incremento dell'occupazione. Ringraziando il

ai presentatori si intendono illustrare le mozioni nn. 77, 86 e 90, già presentate, o se intendano ritirare le stesse a seguito della presentazione dell'ordine del giorno.

Presidente, vorrei dire che noi potevamo comunque illustrare le nostre mozioni, perché facciamo parte tutti dello stesso intergruppo sulla lotta contro il cancro. Perciò, se volevamo esporle, eventualmente potevamo farlo.

Siamo ancora in attesa, ma speriamo che il Registro nazionale tumori venga al più presto attuato, perché credo che possa diventare

un male come questo, la prima sensazione è quella di solitudine e di ricerca di una soluzione veloce, che possa dare comunque speranza, anche se non

In tutti questi anni abbiamo sentito storie di coraggio e di vittoria da parte delle donne e dei grandi passi in avanti che sono fatti per la cura del tumore al seno.

delle nostre università e dei nostri istituti ospedalieri. Mi piace chiudere pensando che la ricerca vada supportata, ma soprattutto finanziata, più di quanto è stato fatto finora, perché i ricercatori e gli scienziati che ci sono nel mondo spesso e volentieri non hanno solo un cognome italiano, ma sono italiani. Credo che questo vada ricordato e vada messa in atto una politica seria nei confronti della ricerca a tutto tondo.

l'aspetto pediatrico è di fondamentale importanza e sarebbe un bel segnale, sotto l'aspetto dei finanziamenti nei confronti di questi reparti, porvi attenzione; mi riferisco anche alla strutturazione dei reparti che devono essere a misura di bambino.

Signor Presidente, colleghi, innanzitutto siamo soddisfatti che si sia arrivati su questo tema a un ordine del giorno comune. Ci tengo solo a ribadire che il 7 febbraio 2018 l'Associazione salute donna, assieme a tutte le 23 associazioni che fanno parte di questa rete

nell'ordine del giorno. È stato aggiunto il tema del *caregiver* oncologico, che non era inserito nella mozione originaria, ma i punti più importanti sono: la formazione di un nuovo piano oncologico nazionale, basato sulla centralità del paziente e del suo percorso terapeutico; le reti oncologiche ed ematologiche regionali, a cui bisogna dare attuazione in collegamento anche con il registro tumori nazionale; la messa a punto e l'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali (i famosi PDTA per le diverse forme di cancro); l'accesso permanente delle associazioni dei pazienti presso i tavoli istituzionali, perché non dimentichiamoci che questo associazioni fanno tantissimo per i pazienti e aiutano, anche negli ospedali, a a fare in modo che il paziente si trovi più a suo agio e riesca a superare meglio anche l'aspetto psicologico. Quindi, hanno un ruolo fondamentale e in alcuni casi fanno anche di più. L'altro impegno è mantenere un adeguato e sostenibile finanziamento del Fondo per i farmaci oncologici innovativi. Su questo fronte abbiamo visto in più di un'occasione come il lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici, proprio con metodi innovativi,

per promuovere l'adesione agli *screening* oncologici previsti e garantiti dai Livelli essenziali di assistenza. Questi sono i punti programmatici che tutti condividono costituiscono il percorso ideale per la presa in carico e la cura del paziente oncologico, com'è stato detto anche dal collega che mi ha preceduto. Sottolineo il contributo importante del mondo del volontariato e della società civile a dare uno stimolo su tematiche che non hanno la risonanza mediatica che spesso i politici cercano:

c'è l'idea di proseguire. Auspichiamo quindi che il Governo cominci con qualche atto concreto a venire incontro a queste esigenze, che sono assolutamente importanti.

Signor Presidente, mi scuso con il presidente Romeo per essere stata disattenta nel non considerare la mozione; purtroppo credo che questa disattenzione l'abbiamo avuta in molti senatori,

possa essere tenuta sotto controllo, attraverso un lavoro e un approccio che coinvolgano il Servizio sanitario nazionale. Si tratta di una sfida che riguarda da vicino la politica.

che nasce appunto dall'accordo tra le 21 associazioni di pazienti oncologici del progetto «La Salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere». un Intergruppo costituito da tutti i parlamentari che ha tra gli obiettivi principali l'azzeramento delle notevoli disparità di trattamento dovute purtroppo alle diverse gestioni all'interno delle singole Regioni, che determinano tempi e qualità delle prestazioni profondamente diversi, come tutti purtroppo sappiamo. Nella nostra mozione ricordiamo alcuni punti che oggi terrei a sottolineare. Innanzitutto il finanziamento per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici; noi chiediamo espressamente di garantire la copertura finanziaria

Un altro punto importante per noi è facilitare l'accesso tempestivo dei malati all'innovazione di diagnosi e terapia, superando le disparità esistenti tra i Paesi europei. garantire una copertura finanziaria alle terapie geniche attraverso modelli di finanziamento, sempre a medio e lungo periodo, con vincolo di destinazione. Solo così si potrà

Un punto importante, che chiedo possa essere inserito all'ordine del giorno che condivideremo, è volto ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di disposizioni per la piena integrazione della figura del *caregiver* familiare nell'ordinamento giuridico, riconoscendo la specificità del *caregiver* oncologico e attivando la rete delle cure palliative a domicilio senza inutili attese ed eccessive burocrazie. Si tratta di un punto importante. Gli altri punti sono già stati sottolineati, ma ricordo che

e questo deve essere importante per noi. Abbiamo avuto dei ricercatori di fama mondiale, uno su tutti il professor Veronesi, che ci ha lasciato protocolli fondamentali soprattutto per il tumore al seno.

quello della psiconcologia, una materia sviluppatasi negli anni, che coglie anche l'aspetto psichico di chi è affetto da una patologia oncologica, che deve essere sostenuto. Non c'è solo la parte organica e non dobbiamo curare solo il corpo, ma dobbiamo curare il paziente in maniera

poi diffondere informazioni chiare e puntuali sulla ricerca clinica e facilitare l'accesso agli studi clinici da parte dei pazienti oncologici ed oncoematologici, sempre con l'obiettivo di favorire l'approvazione e la disponibilità tempestiva delle terapie più innovative.

Aderendo profondamente al ragionamento che nasce dal rapporto con le associazioni di volontariato e i familiari, vorrei solo fare una sottolineatura, soprattutto per il Governo. Tutto ciò che affermiamo nell'ordine del giorno e che era sostanzialmente ripreso nelle tre mozioni, che personalmente condividevo, prende atto di un problema oggettivo: la profonda diversità e disparità sul territorio nazionale delle pratiche, a cominciare dalla rete oncologica, dai sistemi di integrazione a quelli di assistenza, di assistenza domiciliare o *caregiver.* È una riflessione che non può fermarsi a questa presa d'atto; c'è bisogno

c'è quel problema di ritardo e di cui abbiamo parlato, per costruire le reti oncologiche integrate occorrono investimenti,

di una scelta economica. Noi abbiamo approvato una norma giustissima, che condividiamo tutti, sul registro dei tumori, ma senza un euro.

dobbiamo, però, assumerci una responsabilità. Dobbiamo dare le risorse indispensabili per realizzare quei punti che qui abbiamo indicato, per sostenere la rete di domiciliarizzazione, che considero fino ai malati terminali. Tenete conto che abbiamo ancora un problema serissimo per quello che riguarda la rete degli *hospice*, perché alcune Regioni sono in grado di rispondere sugli *hospice* ma tante altre Regioni non lo sono. E noi sappiamo che gli *hospice* sono un elemento di civiltà. benissimo questo ordine del giorno unitario, ma troviamo un modo, signor Sottosegretario, per costruire una strategia, per metterci delle risorse, per fare degli interventi concreti. Diversamente, è sì importante la condivisione ma ci fermiamo qui. Occorre decidere un investimento strategico sulla salute, che non è solo una spesa, ma è un investimento. Noi siamo in recessione. La salute, la sanità, la sanità, sono un grande sistema di investimenti, che può consentire di far crescere questo Paese. Smettiamo di ragionare solo come se fosse una spesa. Abbiamo aziende farmaceutiche importanti in questo Paese. Dobbiamo gestire la grande sfida dei farmaci innovativi, che ci propone di cambiare le norme sui farmaci maturi per gestire il tema dei farmaci innovativi. Bisogna fare delle scelte.

Signor Presidente, stimati senatori, non posso che essere felice di questa condivisione, veramente bella, da parte di tutte le parti politiche. ne sono felice sia come rappresentante del Governo che come addetto ai lavori, visto che ho speso trentacinque anni della mia vita nella ricerca oncologica. Quindi, questo è un momento di gioia per me. per me. Chiaramente è tutto condivisibile, soprattutto quest'ultimo intervento del senatore Errani. Io auspico che continueremo con questo passo, come già fatto per il registro tumori, già fatto per la rete degli IRCCS. Per quanto concerne le campagne di prevenzione, esistono effettivamente, ancora oggi, differenze sostanziali tra Nord e Sud Italia. Questa è una realtà e il Governo si impegna, e particolarmente mi impegno io, visto che ho la delega specifica per queste problematiche, a fare del mio meglio per cercare di sanare queste differenze. Credo che il cancro sia un problema che riguardi chiaramente tutti e, quindi, io auspico, anche nel prossimo futuro, di trovare sempre un allineamento completo da parte di tutte le forze politiche per sostenere questo tipo di attività, sia per la prevenzione, sia per la diagnosi sia per le terapie. Oggi le terapie innovative sono una sfida importante. Volevo qui approfittare solo per fare un po' di chiarezza tecnica - consentitemelo - su alcune terminologie. La terapia genica è di per sé una piccola parte delle terapie innovative. Ci sono anche terapie molecolari. Quindi, è più appropriato, dal punto di vista tecnico, parlare di *molecular di *molecular target therapy*, terapie di precisione più che terapie personalizzate. Le terapie personalizzate non esistono, sono un ideale. Le terapia di precisione sono quelle terapie

proponendo di apportare comunque un'integrazione in tema di educazione sanitaria. Da cittadino e da medico apprezzo la politica sanitaria che mette sempre al centro il paziente, sia come singolo individuo sia come componente delle associazioni portatrici di interesse, le quali devono sempre essere coinvolte nel dialogo e nel confronto con le istituzioni sanitarie. Mettere al centro il paziente significa - da parte di noi medici - garantire allo stesso una corretta informazione al fine di renderlo consapevole e partecipe motivato delle decisioni che riguardano il proprio benessere e il proprio percorso terapeutico, ove necessario. Mettere al centro il paziente significa ancora prima consentirgli di acquisire una corretta educazione alla salute, la quale costituisce un pilastro fondante del nostro Servizio sanitario nazionale sin dalla sua nascita, con legge n. 833 del 1978. Tale legge, tra le sue finalità, prevede la formazione di una coscienza sanitaria che permetta a ciascun individuo di prendere decisioni consapevoli circa il proprio equilibrio e il proprio benessere fisico, psichico e sociale, vale a dire decisioni in merito alla propria salute. La salute - lo ricordo - secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, non è solo assenza di malattia; è uno stato di benessere fisico, psichico e sociale dell'individuo. Per questi motivi propongo l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione sanitaria nelle scuole come disciplina obbligatoria al fine di accrescere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza della prevenzione delle malattie e dell'adozione di corretti stili di vita. Tale insegnamento dovrebbe comprendere al proprio interno vari ambiti, tra i quali la promozione della dieta mediterranea e dell'attività fisica e la lotta contro l'uso di sostanze dannose come il fumo, l'alcol e le droghe, pratiche e abitudini che riducono il rischio di malattie degenerative e oncologiche. Dovrebbero essere inoltre previste specifiche giornate con visite di istruzione dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute presso le aziende sanitarie e altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché università ed enti di ricerca. Auspico pertanto l'aggiunta, tra le misure per fronteggiare le malattie oncologiche, di un impegno all'ordine del giorno G1 affinché il Governo inserisca l'insegnamento dell'educazione sanitaria nel novero delle discipline obbligatorie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, la mozione presentata da Forza Italia, brillantemente illustrata dalla collega Rizzotti, che ha trovato grande adesione e condivisione, ancor prima del valore politico e di impulso legislativo ed esecutivo, voleva essere la raccolta del grido di allarme e dolore che proviene da chi, ogni giorno, deve combattere contro un male dai contorni oscuri con armi che sono ancora, per troppi versi sconosciute. Inoltre, la mozione voleva dare risposte concrete ed efficaci alle famiglie che devono combattere contro il cancro. Colleghi, il cancro, purtroppo, ancora oggi, è un male di cui non conosciamo l'eziologia precisa e miete moltissime vittime ogni anno. In un recente passato, l'essere ammalato di tumore ingenerava la massima solidarietà, considerando - per un verso - l'elevata mortalità della patologia e - per altro verso - l'eccezionalità dei casi. Oggi, invece, assistiamo a una tragica diffusione del male che non conosce età, confini geografici, latitudini e razza. Nonostante siamo in presenza di un male così grave e invalidante tanto per gli ammalati, quanto per le famiglie la risposta che il nostro Servizio sanitario nazionale fornisce è, per alcuni versi, assolutamente insoddisfacente.

che riesca a combattere il cancro con tutte le armi possibili a nostra disposizione: piano oncologico nazionale, reti oncologiche regionali e applicazione reale dei costi *standard*, fino ad arrivare di campagne di sensibilizzazione per potenziare in tutto il territorio nazionale gli *screening* oncologici garantiti dai livelli essenziali di assistenza.

in tutti i settori - in particolare nella materia sanitaria - siamo felici che in una materia così delicata, che riguarda la salute di tutti i cittadini, si sia trovato un importante accordo che ha consentito di approdare alla massima condivisione possibile dell'ordine del giorno, di modo che il Governo potrà impegnarsi da subito per migliorare le aspettative di vita e le condizioni di cura dei malati oncologici. Di fronte a un nemico comune come il cancro non ci possono essere divisioni, ma si deve marciare tutti uniti fino alla meta che consentirà, nei prossimi anni, di considerare il tumore un male sempre più curabile e, nei prossimi decenni, di eliminarlo dalle nostre vite. Forza Italia rimarrà vigile anche con riferimento a quanto abbiamo appena chiesto ai colleghi della Lega, utilizzando tutti gli strumenti politici necessari

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è disamina di un qualunque dato nel nostro Paese che non ci porti a constatare che esistono, purtroppo, differenze sostanziali da area ad area e da Regione a Regione nell'approccio alla programmazione e alla pianificazione in tutti i settori strategici. Tali divergenze risultano assolutamente non degne di uno Stato civile, soprattutto quando hanno a che fare con cure, terapie e assistenza in campo sanitario. È da quando abbiamo messo piede in quest'Aula che abbiamo assunto un impegno, ovvero fare in modo che la sopravvivenza e la salute di un qualunque cittadino non debbano mai più dipendere dal luogo in cui è nato. Ci siamo battuti fin da subito perché l'Italia si potesse dotare finalmente di una Rete nazionale dei registri dei tumori, in grado di consentire l'approccio alle migliori terapie, tenendo conto di dati oggettivi su fattori di incidenza e prevalenza di patologie in rapporto a determinate aree geografiche, raccolti su tutto il territorio nazionale e fatti confluire su un'unica piattaforma. L'impegno che chiediamo oggi al nostro Governo è di ridurre, fino a cancellarlo del tutto, il *gap* tra alcune Regioni provocato dalla disparità nell'approccio al trattamento delle patologie tumorali. Un ragionamento che va affrontato a partire dalla prevenzione, che necessita di campagne e strategie di comunicazione che stimolino ed incentivino le comunità ad affrontare gli *screening* oncologici che rientrano nell'offerta dei livelli essenziali di assistenza, fino alla presa in carico del paziente, che determina la qualità del percorso terapeutico. Il nostro riferimento deve essere la risoluzione di maggio 2017, emersa dalla settantesima Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità, sulla prevenzione ed il controllo del cancro. Con quel documento gli Stati membri si sono impegnati a definire i rispettivi piani nazionali di controllo del cancro, a cominciare da una migliore qualità di raccolta dati ai fini dell'implementazione dei registri, promozione della prevenzione e all'attivazione di ulteriori piani di riduzione del fumo. La stessa risoluzione raccomanda, inoltre, di porre in essere attività rivolte alla diagnosi precoce di sviluppare protocolli diagnostico-terapeutici e assistenziali rivolti alla gestione della patologia; di promuovere un ricorso sostenibile agli strumenti di diagnosi e cura dei tumori; di assicurare ai pazienti, laddove necessarie, le cure palliative; di promuovere la ricerca sul cancro; di favorire forme di collaborazione fra le autorità e le associazioni di pazienti e l'impiego del *counseling* psicologico. È un dato di fatto che i passi in avanti compiuti nell'ambito delle terapie poco o mal si coniugano con l'accesso alle stesse. La maggiore criticità, in questo senso, è costituita dall'eccessiva frammentazione delle decisioni a livello territoriale.

Senza riprendere gli impegni già ricordati dai colleghi, dal senatore Romeo e dalla senatrice Boldrini, voglio aggiungere che l'ordine del giorno G1 impegna il Governo a dare effettiva attuazione alle reti oncologiche ed ematologiche regionali ed al registro tumori nazionale. impegna il Governo a favorire l'istituzione nelle Regioni del centro accoglienza e servizi, che deve essere la porta d'ingresso e l'inizio del percorso diagnostico-terapeutico per il paziente oncologico; oncologico; a favorire la diffusione e l'accesso ai *test* diagnostici molecolari che permettono di accedere a terapie *target* personalizzate, utilizzando in modo appropriato le risorse del Servizio sanitario nazionale. Impegniamo altresì il Governo a garantire la corretta informazione del medico al paziente per ottenere una piena condivisione nel caso si opti per uno *shift* terapeutico. Infine, impegniamo il Governo a lavorare per garantire, nel rispetto dei vincoli della sostenibilità del sistema e delle necessità dei pazienti oncologici e oncoematologici un accesso regionale il più rapido possibile alle nuove terapie, anche attraverso sistemi alternativi ai prontuari terapeutici ospedalieri regionali, come già fatto in alcune Regioni. Nel dichiarare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, invito tutti a lavorare insieme per raggiungere una strategia che sia sempre più mirata a ridurre le differenze territoriali e ad adeguare le cure e l'assistenza alle metodologie più all'avanguardia per permettere ad ogni singola Regione di essere in linea con gli approcci terapeutici più innovativi. Non vogliamo più cittadini di serie A e cittadini di serie B. Il nostro Servizio sanitario nazionale resta un modello invidiabile in tutto il mondo. Dobbiamo e possiamo migliorarlo, impegnandoci sempre di più per sanare le disparità tra le diverse aree del Paese nell'accesso a trattamenti fondamentali e ponendo un argine alla migrazione sanitaria, che in certi territori, soprattutto in campo oncologico, sta assumendo caratteri sempre più allarmanti.

Il caso ha voluto che a presiedere ci sia una persona che il cancro lo ha avuto e da sei anni e mezzo lo sta combattendo.

Signor Presidente, le comunico e comunico agli onorevoli colleghi che il Governo ha trasmesso alla Commissione finanze il testo dell'avviso di rettifica inviato in data odierna alla *Gazzetta Ufficiale* relativo al provvedimento al nostro esame.

Comunicato relativo al decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante: «Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. Cassa di risparmio di Genova e Imperia.» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2019). Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, seconda colonna, all'articolo 20,

Signor Presidente, gli errori possono capitare anche nello scrivere una legge. Certo io non ricordo che ci sia stata una modifica a un testo di legge - perché questa è una legge dello Stato, non è un disegno di legge - in vigore dal 9 gennaio scorso, quindi vale la pena andare a vedere come mai c'è stato questo errore. Giova, come mi ha suggerito la senatrice Modena, confrontare il testo del decreto-legge che stiamo esaminando con il testo del decreto-legge n. 237 del 23 dicembre 2016 firmato dal presidente del Consiglio Gentiloni Silveri e dal ministro Padoan, «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio e del settore creditizio». Ebbene, i primi 19 articoli sono, con l'eccezione di due, nella rubrica e in grandissima parte del testo, perfettamente uguali al decreto-legge che stiamo esaminando.

La cosa curiosa è che io allora sono andato a vedere anche i Resoconti. All'epoca l'approvazione non è stata proprio tanto liscia, perché alla Camera il MoVimento 5 Stelle (l'ho ricavato sia dal Resoconto, sia

lavori. Gli amici della Lega hanno esposto cartelli con scritto "risparmiatori truffati",

copia male e credo che voterà a favore.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento a tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario. Lo facciamo nella speranza che Carige trovi un *partner* all'altezza, in particolare per quel che riguarda la salvaguardia dei posti di lavoro. In molti interventi, anche nel dibattito alla Camera, si è parlato delle responsabilità e del sistema dei controlli che, come nel caso delle altre banche, non ha fatto fino in fondo il suo dovere. Mi unisco anch'io agli interrogativi che sono stati sollevati e aggiungo due considerazioni di ordine generale. La prima è che questo provvedimento è un copia e incolla di quelli approvati nella passata legislatura. È la conferma che, quando le situazioni arrivano a un tale livello di criticità, per la politica non c'è altra strada percorribile per scongiurare una crisi del sistema bancario e per tutelare gli interessi e i risparmi di tutti. Chi governa non può fare altrimenti, ma chi può invece scegliere cosa fare sono le opposizioni. Possono strumentalizzare il tema, attaccare il Governo e dire che salva i banchieri con i soldi pubblici; oppure possono fare un discorso di verità al Paese, dicendo che su certi temi l'interesse generale e il senso di responsabilità vengono prima di tutto. Noi oggi facciamo in quest'ultimo modo e lo facciamo anche perché un domani non vogliamo provare imbarazzo a guardare negli occhi i nostri elettori; quell'imbarazzo che spero in tanti stiano provando nell'attuale maggioranza. Ma di questa vicenda c'è anche un altro aspetto degno di nota. Fa un certo effetto ricordare ai sovranisti di quest'Aula che a spingere l'Italia a prendere iniziative per tutelare i clienti di Carige, quindi la gente, sia stata proprio l'Europa, quella sempre raccontata come cattiva e che, invece, anticipa e spinge il Governo a proteggere i suoi cittadini. La propaganda ha gambe all'inizio molto veloci, che poi si dimostrano corte. Quindi ad inseguirla, alla fine, ci perdono tutti e ci perde, in particolare, la qualità e la bontà del dibattito pubblico della democrazia. Il mio auspicio è che questa vicenda possa essere d'insegnamento e che, soprattutto, questo provvedimento aiuti Carige, i suoi lavoratori e i suoi risparmiatori a uscire dalla difficile situazione in cui versano.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi condividiamo questo provvedimento, che voteremo convintamente:

la tempestività con cui il Governo ha assunto questo provvedimento. Detto questo,

è lo stesso assunto dal Governo precedente in relazione a Monte dei Paschi di Siena e via dicendo. È lo stesso e, da questo punto di vista, la propaganda non riuscirà in nessun modo a nascondere questa semplice verità. Dov'è allora l'occasione persa?

che ci consentisse di andare oltre il classico dibattito propagandistico e inefficace, in primo luogo in relazione, per esempio, a che cosa possiamo fare insieme sul piano dell'iniziativa parlamentare per sostenere sottolineo la parola «sostenere» - il Governo nell'intervento di modifica delle norme europee che per il nostro Paese non vanno bene.

Siamo tutti pronti a lavorare per superare il *bail in*? Come facciamo? Costruiamo un'iniziativa insieme. C'è l'attività di indagine

ma lavori per capire invece che cosa possiamo e dobbiamo fare per migliorare e rendere più efficace la normativa, fino a quella sui controlli. Ora, se la può prendere con Banca d'Italia, ma come avete detto anche voi in alcuni interventi interventi le indagini e anche le sentenze su Carige nascono da un'iniziativa assunta da

della democrazia nel nostro Paese. È un fatto molto importante. C'è un altro punto che vorrei sottolineare, nell'occasione persa: forse

Sono d'accordo che non possiamo essere subalterni ai mercati che sbagliano abbondantemente, come abbiamo visto dalla crisi della Lehman Brothers in avanti. Proprio per questo è fondamentale che il Governo italiano non si isoli in Europa in Europa e non perda tempo nel dare le colpe. Voi oggi governate e dovete farvi carico di costruire un sistema di alleanze in Europa che ci aiuti, visto che abbiamo il secondo più grande debito pubblico al mondo, che purtroppo cresce, e visto che siamo in recessione. Serve un sistema di alleanze

giusto il fatto che dobbiamo salvaguardare una banca "territoriale" che ha una funzione fondamentale, ma c'è da governare governare e salvaguardare il lavoro e i dipendenti di quella banca, che non possono essere i pagatori finali di una malagestione che dura da anni e che si è vista anche, di sentenze della magistratura, condannata severamente. Qui il Governo deve fare un'azione di grande attenzione e di governo, appunto, di questo processo di riorganizzazione e ristrutturazione.

Questo è il motivo per cui ci siamo comportati con senso di responsabilità, pur non condividendo in pieno il contenuto del provvedimento: abbiamo accettato anche le lungaggini derivanti dagli errori tecnici su cui ci siamo soffermati; abbiamo presentato emendamenti non a scopo

Quello che ci fa specie e che pertanto vorremmo sottolineare, invitando alla riflessione anche i colleghi degli altri Gruppi, è il fatto che ormai si ritenga quasi scontato che le banche e gli istituti di credito debbano godere di un trattamento diverso e privilegiato rispetto a tutti gli altri sistemi imprenditoriali del Paese. Mi spiego con un esempio molto banale: stiamo discutendo

Questo è evidentemente uno squilibrio e una situazione paradossale che dovremo affrontare prima o poi, perché sicuramente è giusto difendere i risparmiatori, soprattutto se truffati, ma è anche vero che potrebbero esserci distorsioni, nel momento in cui si sa che l'investimento in banca, alla fine, comunque è garantito dallo Stato, mentre quello che si fa come singolo privato e cittadino in un'azienda che produce mobili, automobili o panettoni non dà questa garanzia. Credo sia una distorsione del mercato degli investimenti su cui forse sarebbe stato il caso di riflettere, ma nessuno su questo ha pronunziato una parola soltanto. Ripeterò quanto detto da altri colleghi, perché è semplicemente la verità oggettiva e incontrovertibile: questo è un decreto-legge copia e incolla di quelli precedenti; è inutile che tentiate di negarlo, l'avete fatto in fretta e furia, nottetempo e, ancora una volta, d'urgenza, perché, dopo aver negato che mai sarebbe successo, anche il Governo giallo-verde si è trovato di fronte alla necessità di non far saltare per aria una banca, con tutte le conseguenze del caso. La fretta, purtroppo - e spero soltanto quella, altre ragioni ingiustificabili - vi ha impedito di fare un intervento sistemico, come spesso annunciato, sul settore bancario.

e indipendenza. Pertanto, al netto del giudizio personale sul professore, sia chiaro che non faremo sconti rispetto alle qualifiche che deve avere per ricoprire una carica così delicata in Consob, perché altrimenti partiamo ancora una volta con il piede sbagliato, dopo aver fatto annunzi che andavano in tutt'altra direzione, cioè quella della massima trasparenza e indipendenza.

tra le banche *retail*, le banche ordinarie e le banche di investimento. Questo è all'origine del travisamento della volontà del piccolo risparmiatore, che non è in grado nonostante le norme, i pacchi di carta, le avvertenze degli sportelli bancari, di distinguere tra un investimento ad alto rischio e uno a basso rischio. Dobbiamo separare le finalità delle banche, altrimenti i risparmiatori saranno ancora indotti in errore. Abbiamo presentato emendamenti - lo ripeto ancora una volta - non a carattere ostruzionistico, per tentare di migliorare il testo. Sono stati in gran parte respinti, alcuni addirittura giudicati, in maniera assolutamente ingiustificata, inammissibili. Voglio ricordarli brevemente. Il primo riguardava un codice di natura etica. Forse la parola etica in politica non andrebbe usata; usate allora un aggettivo che vi piace di più, ma c'è da dire che di fronte al fatto che i soldi

alle retribuzioni dei propri *top manager* in linea con il buon senso. Non si possono più vedere situazioni come quelle a cui abbiamo assistito, con *top manager* che guadagnano milioni di euro, hanno buonuscite clamorose ed ingiustificate, stipendi stellari,

che anche le operazioni relative ai *non performing loan*, ai crediti deteriorati, non diventino un'altra occasione di speculazione a favore di agenzie di banche che fanno questo di mestiere. Presidente e colleghi, chi segue la vicenda sa bene che anche la cessione dei crediti deteriorati è diventata occasione di speculazione. Abbiamo chiesto semplicemente che sia riconosciuto un diritto di prelazione, soprattutto per il piccolo risparmiatore, rispetto alle pratiche di *factoring*, cioè alla cessione del credito, che sia consentito al piccolo debitore di saldare il proprio credito con la banca senza essere oggetto di un'ennesima speculazione condotta da chi lucra lucra interessi giganteschi sulla difficoltà delle banche e sulla difficoltà di recuperare il credito. L'ultima richiesta che abbiamo fatto mille volte, che credo sia una riproduzione di richieste avanzate dai colleghi di maggioranza in altre occasioni, seduti su altri banchi,

che sono stati oggetto di favori, anche a sfondo politico da parte delle banche, che le hanno portate in *default* per l'impossibilità di restituire quanto ricevuto. Cosa impedisce allora al Senato della Repubblica di fare non un ordine del giorno

e beneficiare dei contributi pubblici e delle garanzie pubbliche deve rendere pubblico l'elenco. Avete fatto una norma che costringe anche

senza un processo di riforma, di trasparenza, di eticità e di responsabilità. Altrimenti continuiamo e continuate a dare la sensazione che cambiano i Governi, ma il sistema bancario rimane lo stesso: impenetrabile e immodificabile.

il Partito Democratico voterà a favore del decreto-legge Carige, perché il Partito Democratico voterà a favore del decreto-legge Carige, perché la sua rapida approvazione è utile all'Italia. Lo faremo per due ragioni fondamentali: una riguarda le lavoratrici e i lavoratori della banca, i correntisti, le imprese che hanno crediti e la certezza dell'impatto drammatico che avrebbe il fallimento dell'*ex* Cassa di risparmio di Genova e Imperia sulla Liguria, dove è concentrata gran parte dell'attività della banca. L'altra ragione è la stabilità finanziaria dell'Italia, la tutela del risparmio delle famiglie e la consapevolezza che l'insolvenza di un'importante banca danneggerebbe l'economia nazionale, già alle prese con il rallentamento dell'economia mondiale, proprio mentre il calo della produzione industriale ci porta dentro una vera e propria recessione. All'inizio della XVII legislatura, all'indomani della crisi economica più lunga e profonda dal dopoguerra, ci si è dovuti misurare con le difficoltà specifiche di singoli istituti bancari, frutto anche di errori manageriali. Ci si è dovuti confrontare con la necessità di migliorare la capitalizzazione e la qualità degli attivi delle banche e di rafforzarne la *governance*, nel quadro dell'introduzione della vigilanza unica e nel nuovo quadro dell'Accordo Si è quindi messa in campo una strategia organica di intervento nel settore finanziario, con l'adozione di riforme incisive, mentre in parallelo si gestivano specifiche crisi bancarie, in assenza, inizialmente, di adeguati strumenti. Parto da qui, da questo giudizio netto su quanto fatto dai Governi della scorsa legislatura, che rivendico e rivendichiamo. Voglio qui ricordare il ministro Tria, in audizione, ha ammesso di aver fatto, con il decreto-legge in esame, la stessa cosa dei Governi precedenti, perché è l'unica cosa giusta e possibile che si può e si deve fare in questi casi. se un «fatto specifico è simile a un altro, la norma è la stessa e il decreto è uguale» a quello fatto dei Governi precedenti. «Non vedo come si possa fare un decreto in modo diverso»: così parlò Tria *(Applausi del Governo formato da Lega e MoVimento 5 Stelle. Quindi salutiamo positivamente il fatto che le forze politiche che attualmente governano il Paese abbiano finalmente fatto un bagno di realtà.

non occorre che dica altro. Mi dispiace, signor Sottosegretario, che lei non fosse presente: sarebbe stato veramente pedagogico ascoltare l'illustrazione del senatore Malan.

Mi sono un po' persa, invece, sul tono della replica odierna, in cui ad un certo punto ho sentito parlare di un'ossequiosità che ci sarebbe stata, da parte dei Governi precedenti, nei confronti dell'Europa. Vede, senatore Bagnai, non è molto utile, per contare in Europa, battere i pugni davanti alle telecamere italiane per far vedere che si conta. In realtà le battaglie si fanno ai tavoli giusti ed è molto più utile farle con determinazione lì, che non ostentarle a favore di telecamere in Italia. Quindi salutiamo positivamente il fatto che le forze politiche che governano attualmente il Paese siano arrivate a vedere la realtà, ma non possiamo dimenticare che, nella scorsa legislatura, su decreti analoghi, soprattutto il MoVimento 5 Stelle, ma anche la Lega, abbiano non solo votato contro, ma addirittura presentato eccezioni di costituzionalità. Lo hanno ricordato gli ottimi interventi dei miei colleghi senatori Comincini, Grimani e D'Alfonso. Tuttavia, se oltre al criterio di realtà ci fosse anche una conversione ad una nuova civiltà politica, avremmo ascoltato delle scuse per la vergognosa strumentalizzazione sui decreti banche che è stata fatta nella scorsa legislatura.

devo dire mi ha lasciato costernata: un intervento inutilmente provocatorio, tutto guardando al passato, senza tener conto del provvedimento attuale e neanche del fatto che stiamo parlando di un decreto-legge

anche io lo penso, ma credo che anche il Governo, quando viene in quest'Aula, dovrebbe rispettare con molta più attenzione le forze politiche che rappresentano l'opposizione. PD)*. Tornando al decreto-legge, riteniamo doveroso l'intervento di urgenza del Governo su Carige, a valle - bisogna ricordarlo - del commissariamento della Banca centrale europea. Registriamo al riguardo anche una rinnovata preoccupazione internazionale sull'affidabilità e credibilità dell'Italia. Il provvedimento contiene due opzioni diverse sul futuro della banca, che però a nostro avviso è giusto mettere in campo contemporaneamente: la garanzia per le passività di nuova emissione e l'intervento sul capitale, la cosiddetta ricapitalizzazione precauzionale. La garanzia sui *bond senior* è funzionale alla prioritaria ricerca di una soluzione di mercato per Carige. Questa è l'opzione migliore, che meno impegna risorse pubbliche e più valorizza il patrimonio della banca.

il presidente Conte ha ribadito in Europa lo stesso concetto, ma diverse e destabilizzanti erano state le dichiarazioni dei dioscuri del Governo, in particolare del vice *premier* Di Maio, che inopinatamente aveva parlato di nazionalizzazione della banca, affiancando a ciò anche attacchi contro la Banca d'Italia, che indeboliscono il Paese in un negoziato difficile e dall'esito non scontato. Noi riteniamo positivo che, dopo la conversione del decreto-legge con un ampio concorso delle forze politiche, si possa dire che il Parlamento auspica la soluzione di mercato per Banca Carige, facendo attenzione a quegli errori di mercato a cui ha fatto riferimento il senatore Bagnai e ripresi dall'intervento del collega Non è però in contrasto con quest'obiettivo la predisposizione di una possibile ricapitalizzazione precauzionale, che consenta il contemporaneo ingresso dello Stato nel capitale della banca. Ancorché onerosa, la ricapitalizzazione è ciò che consente di rendere chiaro, a chi fosse interessato ad un'acquisizione di Carige, che non si può negoziare all'infinito contando sull'ulteriore indebolimento della banca. In tal caso, infatti, ci sarebbe l'intervento statale per evitare il fallimento. La successiva collocazione avverrebbe comunque a valori di mercato, poiché la ricapitalizzazione precauzionale ha comunque carattere provvisorio, proprio come nel caso del Monte dei Paschi di Siena. Si tratta di una soluzione di ultima istanza, che noi non invochiamo né auspichiamo, ma che, se si rivelasse necessaria, non dovrebbe essere ostacolata dal Meccanismo unico di vigilanza e dalla Commissione europea sulla base di interpretazioni restrittive e improprie della direttiva sul risanamento sul risanamento e la risoluzione delle banche e della comunicazione sugli aiuti di Stato del 2013. Al riguardo, sarebbe bene che il Governo, invece che isolarsi attaccando Paesi come la Francia, che in questo campo possono avere interessi simili ai nostri, si attrezzasse per un difficile negoziato in Europa che, come sempre accade, richiede capacità di fare alleanze alleanze e credibilità verso gli interlocutori. La BCE ha commissariato Banca Carige con un provvedimento d'urgenza, che probabilmente sconta anche il calo di credibilità che questo Governo ha determinato in questi mesi, che già abbiamo pagato con l'aumento dello *spread* e dei tassi di interesse. Chi ha a cuore il destino di Carige, per quel che rappresenta per la Liguria, per i posti di lavoro, per le imprese e i risparmiatori e per gli stessi azionisti, si deve preoccupare in questo momento di unire e non di dividere, con l'obiettivo primario della tutela della stabilità finanziaria e del risparmio nazionale, da perseguire anche attraverso un confronto costruttivo con le istituzioni Ciò perché è proprio grazie al dialogo portato avanti dai precedenti Governi che l'Italia ha ottenuto quella flessibilità nell'applicazione delle regole europee sulla gestione delle crisi bancarie che ha consentito gli interventi su Monte dei Paschi di Siena e sulle banche venete e che oggi è alla base del decreto-legge Consideriamo questo decreto-legge in totale continuità politica con le scelte fatte negli anni passati, non solo perché si muove nello stesso quadro normativo, ma anche perché sembra andare nella stessa direzione, cioè quella di favorire aggregazioni e acquisizioni che rafforzino la solidità del sistema. Concludo, signor ricordando che Genova e la Liguria stanno vivendo un momento molto difficile dopo il crollo del ponte Morandi perché, nonostante il desiderio e la forza che la città sta dimostrando nel reagire, l'impatto economico di quel crollo ha effetti significativi e importanti sulle attività economiche della città e della Regione. voglio anch'io sottolineare come il piano industriale presentato sia un piano che prevede tagli draconiani sul personale e anche sugli sportelli. Quindi, invito il Governo a seguire con attenzione questa partita, che sarebbe un altro colpo ad una città e a lavoratori che sono in difficoltà. Tenendo conto di queste valutazioni, noi voteremo a favore. E voteremo a favore anche perché, per il Partito Democratico, indipendentemente dalla collocazione in maggioranza o all'opposizione, prevale l'interesse dell'Italia e l'interesse complessivo, in questo caso, della stabilità finanziaria.

Signor Presidente, scusandomi se tolgo un minimo di *pathos* e di *suspense*, esordirò dicendo che, naturalmente, il Gruppo Lega-Salvini Premier-PSd'Az, voterà convintamente in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame e questo non per una particolare subalternità al Governo, ma perché è convinto che sia effettivamente la scelta giusta da fare in questo momento, come è stato ricordato da tutti i colleghi. quindi, potrei anche concludere qui, con una economicità estrema di tempi. Però, siccome sono un keynesiano, permettetemi di espandermi un po' e di fare qualche considerazione. In effetti, questa era una scelta che le circostanze hanno reso obbligata e, quindi, anche il dibattito non ha potuto indugiare tanto sul merito della scelta, ma si è elevato, ha volato alto e ho visto qui delle cose che non mi aspettavo avrei mai visto in vita mia; cose che i miei occhi di umano ancora hanno difficoltà a credere e vorrei condividerle con lei, signor Presidente, a partire dall'ultima, la più simpatica. Ho visto un attacco al sovranismo fatto da parte del rappresentante di un Gruppo parlamentare che è così fiero delle sue radici, anzi, *so stolz seiner Wurzeln*, che è abbastanza paradossale: un Gruppo, che così tanto difende la propria piccola Regione, che merita di essere difesa, perché se la prende con un partito che vuole difendere il suo Paese, che altrettanto merita di essere difeso? Ho visto anche un altro dato paradossale: ci è stata rimproverata la frettolosità. Ho qui un fascicolo di editoriali, che i tempi stretti, giustamente, del Regolamento parlamentare mi impediscono di citare ampiamente, e anche i risultati di qualche ricerca che spiegano come, in ambito finanziario, si debba agire tempestivamente e anche come, in precedenti casi, nel trascinarsi fra Tremonti, Monti, *bonds*, tra il "salviamo così" e il "salviamo colà", intanto il tempo passava e le situazioni si deterioravano. Voi non ci potete rimproverare la fretta. Anzi, ci date un immediato sopravvento, perché ci permettete di rimproverarvi la lentezza, che ha portato certe situazioni a incancrenirsi, fino al punto in cui ora noi dobbiamo gestirle. Ci è anche stato rimproverato di essere inesperti. Devo dire che, in effetti, un altro nodo paradossale è che,

affinché questo decreto-legge fosse la copia esatta di un precedente decreto-legge, mancava uno snodo fondamentale, che tutti ricordiamo: occorrerebbe che il *Premier* annunciasse che è un ottimo affare investire (eccetera, eccetera), come ben ricordiamo. Ora, non voglio dire che non sia un ottimo affare; non faccio valutazioni a mercati aperti. Voglio solo dire, però, che forse dovremmo ricordarci che lì non c'è stata fretta, magari non ci sono stati errori materiali, ma c'è stata lentezza e c'è stato un non completo apprezzamento della gravità della situazione. D'altra parte, colleghi, quando si fece il salvataggio *de cuius*, che qui tante volte è stato citato e rivendicato a modello di quello che questo Governo si trova a fare, venne detto agli obbligazionisti che sarebbero stati tutelati al 100 per cento. Poi, invece, il 31 luglio 2017 si parlò di una conversione in azioni, che allora valevano 8,65 euro, ore ne valgono 1,34: lì le cose sono andate in un modo un po' diverso. Vorrei che ce lo ricordassimo! Quindi, non è andata esattamente così, però questo è il passato e forse dovremmo dimenticarcelo e veramente smettere di rinfacciarcelo, per guardare avanti e per cercare di condividere alcuni principi, senza i quali non riusciremo a rimettere in piedi questo Paese. Avrei due osservazioni da fare, sperando di avere il tempo.

ho statalizzato Carige a mia insaputa: intervenendo in una trasmissione televisiva, ho detto che ritenevo che sarebbe stata possibile una soluzione di mercato. Bagnai nazionalizza. A parte che non sta a me farlo, ragioniamo un po' su questo. Ho apprezzato l'intervento che è stato fatto, in particolare dal senatore D'Alfonso, quando ha auspicato che sia il mercato a produrre soluzioni: il mercato produca soluzioni, diceva diceva in replica alla collega Botto, che aveva espresso un principio, secondo me, fondamentale: quale che sia la soluzione, dovremmo entrare nell'ordine di idee che se lo Stato ci mette i soldi, poi lo Stato gestisce. Questo era il punto. Non è che noi vogliamo nazionalizzare, è che se gli si fanno dei regali o se lo si sussidia,

e questo non ha fatto bene, in tutta evidenza, alla stabilità del sistema finanziario, tanto è vero che siamo qui a intrattenerci con queste tristi vicende, che speriamo arrivino a un punto fermo. Quindi, c'è il problema di decidere insieme quale debba essere il ruolo dello Stato nell'esercizio di quel particolare settore che costituisce il sangue vivo dell'economia di un Paese. Siamo assolutamente sicuri di voler demonizzare la possibile creazione o il possibile potenziamento di un polo pubblico anche in questo settore? Vorrei che ci ricordassimo che il Paese al quale veniamo spesso richiamati ad ispirarci, la Germania, ha il 60 per cento del suo sistema bancario sotto controllo pubblico e oltre 1.500 istituti bancari territoriali, alcuni piccoli, alcuni grandi - qualcuno va male, qualcuno va bene - mentre noi stiamo andando verso una concentrazione estrema. Siamo sicuri che una concentrazione estrema risolva tutta una serie di problemi, inclusi quelli del *moral hazard*, cioè: tante banche *too big to fail* ci risolvono il problema del comportamento irresponsabile del *management*, posto che il problema sia quello? Io non credo, ma queste sono opinioni. Oltre al discorso sul ruolo dello Stato, dovremmo forse chiarirci. È stata spesso evocata - con toni,

A parte che autonomia e indipendenza sono due cose diverse, così come lo sono indipendenza e irresponsabilità e forse dovremmo apprezzare la ricchezza di sfumature del linguaggio italiano che qui dobbiamo parlare, perché quello che si cerca, forse, non è indipendenza,

voglio sentire un rappresentante degli italiani che, qui dentro, dice che gli italiani non si meritano un modello di *governance* come quello della Bundesbank tedesca perché loro non saprebbero come gestirlo. Vogliamo metterci in questa *impasse*? Sono molto curioso di vedere chi avrà il coraggio di dirlo!

Grazie, Presidente. 1, che ci perviene in seconda lettura, in quanto già approvato dalla Camera dei deputati con una sola modifica al testo originario,

la Liguria - ma con rilevanza non marginale sia in Lombardia, che nel Lazio. Questi aiuti, previsti dall'articolo 1 (garanzia per 3 miliardi di euro) e dall'articolo 12 (aumento del capitale a beneficio di terzi) tendono a far sì che Carige - lo ripeto - continui a esercitare la sua funzione, *rectius* - come già detto - che sopravviva. Nel provvedimento e nei suoi allegati non un rigo però è stato speso per la disamina della posizione fiscale di Carige, salvo confermare che a essa competono ben 1,2 miliardi di euro per crediti d'imposta. Sono essi pienamente utilizzabili? E il supero con il reddito imponibile (ignoto) può essere ceduto? Carige, inoltre, tra i suoi attivi - pochi annovera una partecipazione del 4 per cento in Banca d'Italia. Ma che senso ha? Perché non è stata dismessa? Il provvedimento ricalca a larghe linee quelli già visti per Banca Etruria, Banca Marche *et similia*. prevede, con maggiore valenza - lo sottolineo - rispetto alle precedenti indicate norme, l'ipotesi che gli oneri a carico del MEF siano di natura transitoria e che potranno essere azzerati, addirittura, con un interesse anche se minimo, dalla prosecuzione delle attività che si spera porterà nei prossimi anni ad un incremento significativo del valore di Banca ma anche ad utili che le consentiranno di uscire dall'*impasse* e restituire i prestiti ottenuti. Inutile rimarcare che tutte le operazioni gestite dal MEF, con la supervisione di Banca d'Italia, saranno oggetto di accurato esame anche da parte della della Banca centrale europea che, come noto, ha emesso nel gennaio scorso il provvedimento di amministrazione straordinaria. Per quanto concerne le cause del dissesto, mi sembra di poter affermare che la prima, per importanza, non è quella determinata dal periodo di recessione mondiale e nazionale iniziato alcuni anni e che ha comportato sicuramente la riduzione dei depositi da parte dei correntisti e di affidamenti sicuri e profittevoli. Il dissesto, sempre a mio avviso, anche sulla base delle dichiarazioni degli auditi, trae origine principalmente dalla *mala gestio* dell'azienda, con le solite consuete operazioni di concessione di crediti (anche milionari) compiacenti, vale a dire con scarse o nulle garanzie e con l'effettuazione di operazioni a rischio elevato che si sono concluse, purtroppo, nel peggior modo. Gli impegni innanzi indicati devono sì consentire la piena continuità dell'azienda, ma, fatto questo più significativo, evitare perdite per i correntisti e che la mancanza di liquidità provochi, di riflesso, un effetto negativo a carico soprattutto delle piccole e medie imprese, che si vedrebbero costrette ad una stasi che potrebbe portare alla cessazione delle attività con gravi ripercussioni anche sul tasso di disoccupazione. Per tutti questi motivi, soprattutto per gli ultimi indicati, Forza Italia voterà, così come fatto in Commissione, a favore del provvedimento.

abbiamo affrontato in quest'Aula il decreto Carige, provvedimento che punta a tutelare una banca per troppo tempo lasciata in balia degli effetti della crisi finanziaria e di gestioni passate a dir poco avventurose, per usare un eufemismo. Un caso a cui si deve porre rimedio tempestivamente. Voglio focalizzare il mio intervento su un punto in particolare. Intendo cioè chiarire il distinguo tra questo nostro provvedimento e quello adottato dai Governi Renzi-Gentiloni Silveri, giacché in più circostanze, come anche durante i lavori in Commissione, si tende ad affermare che l'uno è la riproduzione anastatica dell'altro. Ritengo necessario chiarire la sostanziale differenza nel *modus operandi* con finalità completamente diverse, poiché è del tutto scorretto e fuorviante paragonare il decreto Carige con il precedente provvedimento. La differenza sarà ancora più netta dopo che la Commissione d'inchiesta sulle banche sarà costituita. Voglio inoltre ricordare il percorso dell'allora neopresidente del Consiglio Gentiloni Silveri, che in breve tempo approvò il provvedimento per autorizzare l'assegnazione di 20 miliardi in favore delle banche in difficoltà. Non solo per Monte dei Paschi di Siena, ma all'occorrenza anche Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Successivamente, la Commissione presieduta da Casini non trovò colpevoli e sapete perché? Perché il 31 dicembre 2017 Monte dei Paschi dichiarò di vantare crediti per circa 10 milioni nei confronti di tredici partiti politici e per 67 milioni nei confronti di persone fisiche che occupavano importanti cariche pubbliche. Invece, con il decreto-legge in esame offriamo garanzie pubbliche su emissioni obbligazionarie di Carige e prevediamo la ricapitalizzazione cosiddetta precauzionale, da considerare come ipotesi residuale a valle della quale, se concretizzata, lo Stato entrerà dentro la banca, senza cederla a prezzo simbolico come è successo in passato per due banche venete e per le quattro banche dell'Italia centrale. Inoltre, con il fondo risparmiatori tuteliamo i truffati, i clienti che hanno avuto fiducia in questa banca ma non sono stati ripagati. Abbiamo istituito un fondo per il ristoro dei risparmiatori italiani di un miliardo e mezzo di euro. Il popolo italiano è un popolo di risparmiatori, lo testimoniano l'alto livello di risparmio delle famiglie, che fa ancora oggi molta gola agli operatori esteri, e il fatto che la maggior parte delle famiglie è proprietaria della casa in cui vive. Quindi, un fondo di 15 volte superiore a quello del Governo Renzi-Gentiloni Silveri, il fondo Baretta, dal nome dell'allora Sottosegretario, che stanziava appena 100 milioni di euro in quattro anni, ossia 25 milioni di euro l'anno, insomma un'autentica elemosina. I cittadini sono stati lasciati da soli, dov'era lo Stato? Questo Governo (e il Parlamento) interviene per tutelare i cittadini e non ha ancora sborsato un solo centesimo. Vero è che all'opposizione non resta altro, per attaccarci, che dire che noi siamo come loro. Lo fanno in ogni modo e ad ogni occasione e non certo per disistima nei loro confronti o per sovrastima nei nostri confronti, lo fanno per confondere artatamente le idee ai cittadini. Inoltre, preciso che sempre grazie a noi anche gli azionisti verranno risarciti. Rilevare la responsabilità penale delle precedenti gestioni bancarie è sicuramente di competenza della magistratura, ma è pure giusto costituire una Commissione *ad hoc* per far emergere la responsabilità politica della vicenda, perché sia chiaro che oltre alla crisi finanziaria anche la cattiva politica ha messo alle corde tanto Monte dei Paschi di Siena quanto Carige. Ricordo che quando nel 2008 è scoppiata la crisi finanziaria, è diventato palese che molti, troppi attori hanno scaricato il problema su Carige. Entrambe le banche hanno legato la loro reputazione alle rispettive città, Siena e Genova, e non sarebbe strano se si costituissero parte civile in un processo per danni di immagine. Il problema dunque non è rappresentato soltanto dal Berneschi, condannato a otto anni e a cui peraltro spetta risarcire 26 milioni di euro. Il problema sono anche i crediti deteriorati che la banca è ancora costretta a smaltire. In realtà, attorno al sistema Carige si era venuto a creare un equilibrio di potere non sempre limpido e che di fatto ha governato il consiglio di amministrazione durante decenni in cui spopolavano la Democrazia Cristiana, i Democratici di sinistra e Forza Italia. Bisogna che i cittadini sappiano finalmente cosa è successo in quella perversa triangolazione tra Berneschi, Burlando e Scajola, fratello del Ministro, legato alla *mala gestio*. Non ci si è accorti o si è fatto finta di non vedere i troppi finanziamenti erogati da Carige senza le dovute garanzie agli amici degli amici, alle solite cordate e consorterie. come non accorgersi della truffa continuata nel tempo e rilevata dalla Guardia di finanza in merito all'acquisto di beni immobili da parte del ramo assicurativo dell'istituto bancario a prezzi gonfiati per reinvestire le plusvalenze all'estero, affare che avrebbe fruttato al solo Berneschi 22 milioni di euro. Presidente, concludo con l'auspicio che la Commissione di inchiesta bancaria di imminente istituzione faccia chiarezza sul caso, individuandone le responsabilità politiche parallelamente all'ottimo lavoro che sta compiendo la magistratura, così come, allo stesso tempo, che il nostro Governo miri a rinsaldare la fiducia nelle istituzioni, mostrandosi attento al benessere dei cittadini, in perfetta sintonia con l'articolo 47 della Costituzione, che recita: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Pertanto, il Gruppo MoVimento 5 Stelle dichiara voto favorevole. Prima di procedere alla votazione finale, informo l'Assemblea che l'avviso di rettifica del quale ha dato lettura il rappresentante del Governo è pubblicato nella versione *on line* della *Gazzetta Ufficiale* di mercoledì 6 marzo 2019, a partire dalle ore 19

Ahmadreza Djalali, per anni collaboratore dell'Università del Piemonte Orientale (anni durante i quali ha fornito un contributo fondamentale per la nostra ricerca), è rinchiuso in carcere in Iran con sul capo una condanna a morte per l'accusa di spionaggio. Una sentenza pronunciata dopo che in un video, trasmesso dalle TV iraniane, Djalali avrebbe ammesso di essere una spia; una confessione che sarebbe stata estorta sotto torture e minacce di ritorsioni ai danni della moglie e dei figli (tesi sostenuta da sempre dai legali dell'uomo). Prima della sua confessione, Djalali aveva infatti puntualmente e sistematicamente respinto le accuse nei suoi confronti. In una lettera fatta uscire dal carcere e diffusa dalla moglie, aveva rivelato che la sua condanna sarebbe stata nient'altro che l'effetto di una ritorsione per essersi rifiutato di farsi assoldare come spia al servizio del Ministero dell'*intelligence* iraniano. Versione della quale il tribunale di Teheran non ha mai tenuto conto nei due unici gradi di giudizio. Ricercatore specializzato in medicina dei disastri, nato in Iran ma residente in Svezia, Djalali era stato arrestato in occasione della sua ultima visita accademica in Iran, dove si era recato su invito ufficiale dell'università di Teheran. Di lì a pochi giorni lo hanno messo agli arresti per una presunta "collaborazione con un Governo ostile"; secondo l'accusa, avrebbe passato informazioni al Mossad, l'*intelligence* israeliana. Appare oramai chiaro che c'è chi ha voluto che si autoaccusasse pubblicamente, così da poter mostrare al mondo la prova provata di un'attività di spionaggio che non è mai esistita. L'appello che intendo lanciare oggi da questi banchi è rivolto al nostro Governo, affinché l'Italia, Paese che ha avuto l'onore di ospitare Djalali in una delle sue università e beneficiare della sua opera e dei suoi insegnamenti, possa attivarsi per garantire a quest'uomo un processo equo e giusto, al cospetto di un tribunale indipendente e imparziale, che non potrà che portare alla sua liberazione dopo che sia stata finalmente riconosciuta la sua innocenza. Non possiamo più consentire che si continui a perpetrare questa gravissima violazione dei diritti fondamentali di un cittadino e che, nel contempo, sia messa in gioco la libertà di fare ricerca.

*(M5S)*. Signor Presidente, il 24 febbraio scorso si sono tenute, come noto, le elezioni per il rinnovo del Presidente e dell'Assemblea legislativa della Regione Sardegna. Nella sera del 24, a urne chiuse, la terza rete Rai ha trasmesso uno speciale elettorale, nel corso del quale è stato diffuso un risultato di *exit poll* realizzato, per conto della televisione pubblica, da un *pool* di istituti di rilevazione riuniti sotto l'egida del Consorzio Opinio. I risultati sono stati presentati evidenziando che gli stessi erano frutto di un'elaborazione originata da interviste realizzate all'uscita dei seggi. Il dato proposto, per quel che riguarda i candidati a Presidente, si è rivelato lontanissimo dal 3 per cento dato dallo stesso Consorzio Opinio come limite massimo dello scostamento. L'aspetto più grave che voglio qui sottolineare è che questo ha generato un'evidente distorsione del dibattito pubblico, sia nel corso degli speciali televisivi durati fino a tarda notte, sia, complice il ritardo nell'arrivo dei dati reali, per buona parte della mattinata della giornata successiva, incidendo anche sull'orientamento dei titoli di tutti i giornali in edicola nella giornata del 25 febbraio. È appena da ricordare che, da quando esiste l'elezione diretta del Presidente della Regione, non si era mai verificato in Sardegna, come nelle presenti elezioni, un distacco così significativo tra il primo e il secondo arrivato (15 per cento a favore del primo, 100.000 voti in più), mentre gli *exit poll* prevedevano un testa a testa. Al di là del dato specifico e dei partiti favoriti o danneggiati dai macroscopici errori del Consorzio Opinio e considerato che - stando alle notizie di stampa - lo stesso *pool* di istituti viene remunerato dalla Rai attraverso un contratto che prevede il pagamento di 5 milioni di euro per un biennio, con opzione per il terzo anno, sarebbe bene sapere quali indirizzi intenda assumere l'azienda televisiva di Stato per evitare che il servizio pubblico ingeneri distorsioni di questo tipo nel dibattito politico, rendendosi oltretutto protagonista di un evidente spreco di danari

senatrici e senatori, la procura di Firenze ha appena notificato la chiusura delle indagini a 45 professori e ricercatori di diritto tributario per l'inchiesta che nel 2017 portò a sette arresti e all'interdizione dalle università per altre 22 Tra i reati contestati ci sono quelli di induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione; turbata libertà del procedimento di scelta nei concorsi; abuso d'ufficio; frode; truffa e La procura ora, per questi 45, si appresta ad avanzare la richiesta di rinvio a giudizio. L'indagine nacque dalla denuncia di un coraggioso ricercatore tributarista che fu «invitato» a ritirarsi da un concorso. Da questo spaccato gli inquirenti ricostruirono una rete nazionale di relazioni tra società scientifiche dove, secondo l'accusa, venivano illecitamente concordati i vincitori dei concorsi, con lo scambio di favori e abilitazioni alla docenza. Dopo due anni l'università di Firenze è scossa da una nuova inchiesta. Questa volta nell'occhio del ciclone è finita la facoltà di medicina, dopo la denuncia di un professore associato di otorinolaringoiatria. Sono 14 i professori indagati, ai quali si contestano i reati di abuso d'ufficio e turbamento di procedimenti amministrativi, violenza, minaccia o con doni e promesse. Dopo mesi di intercettazioni telefoniche e ambientali, emerge un universo torbido fatto di intrighi ed astuzie, di relazioni sessuali clandestine in corsia, di desideri morbosi di potere, di truffe e mazzette. Le intercettazioni sono simili ad altri casi: «Lui non deve vincere. Questo posto è per un altro», ma «se facciamo un concorso lo vincerebbe lui». Come in molti altri casi, il sistema capisce che il ribelle è diventato ingestibile. Rimane solo, ma con coraggio denuncia. Da questi atti e dalle inchieste lette sui giornali emergono grandi manovre sui concorsi, così da muovere professori e commissioni come pedine su una scacchiera nazionale. È un gioco ad incastri in tutta Italia che interessa molti settori disciplinari, non tutte le università, ma troppe. I casi hanno coinvolto Catania, Messina, Bologna, Roma Tor Vergata, Roma La Sapienza, Chieti-Pescara, Ancona e moltissime altre città. Quanto alle vittime, ringrazio il senatore Astorre per avermi citato per il mio caso personale, ma, al di là di questo, voglio far presente che qui rappresentiamo altre persone e io qui non sono solo Pierpaolo Sileri, sono anche Giulia, Sandro, Gianbattista, Walter, Fulvio, Agnese, Adamo, Paolo e potrei citare altre decine Quanti ricercatori, professori associati e ordinari, funzionari amministrativi, direttori generali di università e di ospedali e direttori di dipartimento dovranno passare davanti a un giudice a rendere testimonianza? Davvero serve una sentenza per affermare che l'università è malata? Quanti altri dovranno denunciare ciò che subiscono, rimanendo poi isolati, deprivati della loro libertà professionale, dei sogni coltivati da studenti, divenendo esempi per i colleghi: non esempi positivi non di coraggio, come dovrebbe essere, ma esempi per dimostrare cosa ti accade se ti ribelli, diffondendo omertà ed arrendevolezza. Quanto tempo dovrà passare prima che queste organizzazioni criminali di colletti bianchi, rette da omertà, da paura e regolate da riti, legami familiari e percorsi particolari di vendette, che impongono la propria volontà con mezzi spesso illeciti per inseguire interessi privati, vengano chiamate con il nome giusto, cioè mafia?

nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, dopo la partita Fiorentina-Atalanta, tra le Forze dell'ordine e i tifosi. Ci sono dinamiche poco chiare che vanno chiarite. C'è un'interrogazione analoga presentata alla Camera: il Ministro scelga a quale Ramo del Parlamento presentarsi, ma venga e chiarisca quello che è successo, perché i cittadini, prima ancora che i tifosi, meritano parole di chiarezza e meritano che venga fatta piena luce su dinamiche tutt'ora non chiare.

oggi per il Comune di Castelfidardo è una giornata di lutto cittadino, dichiarata dal sindaco Ascardi per la tragedia che il 3 marzo ha colpito la sua collettività: un incidente che a Porto Recanati ha privato della vita due coniugi e che poteva e doveva essere evitato. nella sua ordinanza il sindaco descrive la sua collettività come di persone impegnate per il sociale e indica i due coniugi come il meglio di quella collettività. Io sono testimone diretto della veridicità della sua dichiarazione, perché ricordo perfettamente che quando il mio Comune ha avuto bisogno di aiuto, dopo lo sciame sismico che ci ha colpito nel 2016, il Comune di Castelfidardo è prontamente intervenuto, appunto, per portare solidarietà concreta. Ovviamente per i due coniugi non possiamo fare nulla; potremmo però e dovremmo fare qualcosa per i loro figli. Potremmo e dovremmo fare qualcosa per tutti noi, perché come diceva una famosa canzone tanti anni fa «gli altri siamo noi» e quello che è successo a una famiglia che tornava da una bella serata con gli amici potrebbe accadere a tutti noi, se non arriveremo a disciplinare un problema che purtroppo riguarda tutta Italia. È per questo che,

per far sì che queste assurde tragedie possano essere ridotte, se non addirittura eliminate. *(Applausi